un termine che dovrebbe esservi molto caro, perché non passa giorno che non veniamo chiamati nelle Aule parlamentari per esprimere un voto di fiducia o, per quanto mi riguarda, orgogliosamente di sfiducia.

*partner*, Matteo Renzi, risuonino nei vostri cervelli in modo molto forte. La fiducia non esiste realmente neanche tra di voi, ma, contando sul potere delle poltrone, venite a chiederla giornalmente, in Aula. Su cosa dunque, la fiducia? Su una manovra che, nel giorno della vigilia di Natale, uno dei principali giornali economici nazionali, «Italia Oggi», ha definito «manovra mille e una mancia». È su questa legge di bilancio che voi volete la fiducia? Probabilmente la raccoglierete, colleghi, tra poco più di un paio d'ore. La raccoglierete per quelle ragioni che gli italiani hanno ben note, ma quando sarà il momento sapranno certamente farvi scontare questa vocazione alla poltrona e al potere a dispetto della volontà nazionale. una manovra - ve lo dimostrerò - fatta di mance e mancette; una manovra da 40 miliardi che si aggiungono agli oltre 100 miliardi dei decreti Covid che hanno indebitato questo Paese, hanno indebitato noi, i nostri figli e i nostri nipoti. Ma non lo avete fatto, come avrebbe richiesto l'emergenza, per riforme strutturali e per una manovra davvero straordinaria, come straordinaria doveva essere in un momento così delicato per il nostro Paese. Lo avete fatto per elargizioni, mance e per altri motivi che adesso andremo ad elencare. Serviva invece una manovra rivoluzionaria e straordinaria, come straordinari sono i tempi che stiamo vivendo; una manovra che desse finalmente al nostro Paese quelle riforme nel campo fiscale, della giustizia e della sanità che tutti invocano da anni, da ogni parte politica ed economica. Se non si fanno queste riforme, se non si cerca almeno di impostare queste riforme, quando si spendono 140-150 miliardi in pochi mesi, quando pensate che questo Paese possa davvero avviare il ciclo delle riforme necessarie al nostro futuro? Probabilmente a voi, cari colleghi del Partito Democratico, interessava di più, in questo momento, mettere a posto Monte dei Paschi di Siena e UniCredit, come molto correttamente vi ha spiegato il collega Urso ieri. Era più importante sistemare Padoan, sistemare gli interessi privati di una banca, o meglio di due banche, che ora finiscono nell'alveo del vostro potere, non riconosciuto dal Paese ma riconosciuto dalla vostra burocrazia, dai vostri interessi e dai vostri interlocutori di Bruxelles. Quindi, gli amici del MoVimento 5 Stelle (mai lo avrei pensato), pur non condividendo da sempre gran parte delle loro posizioni, si sono resi "strumenti" (voglio usare un termine gentile) perché questo potesse accadere; strumenti per essere da una parte proni agli interessi economici e finanziari dell'alta finanza e, dall'altra, strumenti per essere nuovamente proni ad un'Europa che ci sta irridendo. È la vostra Europa, che non è la nostra, che sta permettendo alla Germania, che ne è il traino, di acquistare milioni di dosi di vaccino a discapito degli altri Paesi europei. Questa è la vostra Europa, questo è il vostro falso europeismo, che è comodo soprattutto a portarsi a casa le banche, ma non a fare gli interessi degli italiani. Diamo allora anche un'occhiata a qualche numero. una manovra che balla. Non mi era rituale, ma ormai lo sto facendo spesso, citare giornali che da sempre vi sono affini. Avete letto «la Repubblica» di oggi titola: «Svolta o perdiamo i fondi Ue»? Cosa vuol dire, tradotto nella lettura della legge di bilancio? Vuol dire che la vostra legge di bilancio, oltre ad essere politicamente inconsistente,

delle sovvenzioni europee e dei fondi UE. Voi basate una manovra di 40 miliardi sulla

Quindi, la vostra manovra di bilancio non sta in piedi nei contenuti politici e non sta in piedi nelle coperture finanziarie. mi permetta di ricordare in conclusione che avreste potuto anche fare qualcosa, almeno nella legge di bilancio, per gli invisibili e per i professionisti. Anche ieri Marina Calderone, presidente del Comitato unitario Professioni, vi ha accusato di non riconoscere il ruolo dei professionisti. Non avete fatto nulla, non avete risposto ad alcun grido ad alcuna richiesta politica ed economica di questo Paese. Avete però risposto ai vostri interessi personali e privati, agli interessi di Monte dei Paschi, di Padoan, dell'UniCredit. Gli italiani se lo ricorderanno; prima o poi andremo a votare

Signor Presidente, oggi votiamo il provvedimento cardine della manovra economica che chiude l'anno in corso. Un anno, il 2020, che non ha precedenti nella storia del nostro Paese, segnato dalla grave pandemia da Covid-19, che ha stravolto le vite e il lavoro di tanti italiani. Un anno che ha richiesto a tutti noi, in Parlamento e al Governo, un lavoro straordinario, spinti dall'esigenza di tutelare ogni settore, ogni filiera, ogni singolo lavoratore danneggiato dagli effetti della pandemia e nel frattempo prevedere le misure e gli investimenti per costruire l'Italia del futuro. Tra manovra e decreti emergenziali stiamo iniettando nell'economia oltre 140 miliardi di euro, pari a cinque finanziarie in un solo anno. Si comprende che si tratta di una mole di interventi senza precedenti approvati in tempi assolutamente rapidi. Allo stesso modo abbiamo previsto tantissimi strumenti per risollevare il Paese, senza lasciare indietro nessuno. è breve e non voglio leggere tutto il mio intervento. Vado velocemente e perciò dedico solo pochi minuti ai temi più importanti della manovra, quelli più richiesti dai cittadini: il lavoro e l'occupazione. Vi sono misure importanti in questa manovra sul versante della contribuzione per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda le assunzioni di giovani fino a trentacinque anni, specificamente per quanto riguarda l'occupazione femminile femminile e il soccorso e il sostegno alle imprese che assumono nel Mezzogiorno, la cosiddetta Decontribuzione Sud. mi tocca molto - è stato rafforzato lo strumento "Resto al Sud", ampliando la fascia di età per la presentazione dei progetti. Questi strumenti, uniti all'estensione fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e in attività di ricerca nel Mezzogiorno, uniti al potenziamento dell'incentivo "Occupazione Giovani" al Sud e al potenziamento delle zone economiche speciali (ZES), per permettere a questi territori di avere semplificazioni amministrative e sgravi fiscali esclusivi,

A questo proposito voglio anche evidenziare che investire al Sud non significa privilegiare una parte del Paese, facendovi confluire risorse destinate a rimanere sul posto. Certo che no, perché tra Sud e Centro-Nord vi è una grande interdipendenza economica (lo sappiamo), tanto che, come molte ricerche hanno ormai dimostrato, per ogni 100 euro investiti al Sud si produce a beneficio del Centro-Nord un ritorno di ricchezza addirittura superiore al 40 per cento del valore dell'investimento. Questa tipologia di investimenti è un aiuto concreto a tutti i territori, in particolare a quelli più svantaggiati, una spinta per diminuire la disoccupazione nell'intero Paese, un riequilibrio sociale, un riequilibrio sociale, del quale abbiamo tanto bisogno, e un concreto aiuto a tutto il sistema Paese. Sono previsti altri numerosi e rilevanti temi nella legge di fondamentali per la ripartenza dell'economia che seguirà la pandemia, cogliendo anche l'opportunità che ci offre di preservare l'ambiente di cui siamo parte integrante. Penso soprattutto al grande tema della transizione energetica. Nato come un sogno, ora sta diventando una realtà. Abbiamo incentivato l'acquisto di auto a bassa emissione e reso obbligatorio, per i concessionari stradali, di installare le colonnine di ricarica per auto elettriche di ultima generazione. Abbiamo prorogato il super bonus al 110 per cento, molto atteso, ossia una misura straordinaria per rendere più sicure e più efficienti energeticamente le nostre case. grazie soprattutto al sostegno totale dello Stato. Questa misura viene estesa al 2022 e contiamo di estenderla ancora almeno fino al 2023, per consentire la creazione di un vero circolo virtuoso, capace di creare una spinta *shock*

Vorrei rispondere a qualche critica che è venuta dai banchi dell'opposizione. È vero, come dicono: il provvedimento in esame ha visto l'intervento attivo di una sola Camera. in un anno ordinario, avrebbe significato un grave *vulnus* per il bicameralismo e per la democrazia, ma in quest'anno straordinariamente difficile, segnato dalle emergenze e dalla necessità di fare presto e bene, nell'ottica esclusiva dell'emergenza, l'inedita capacità di collaborazione tra le due Camere, che, di fatto, hanno fatto convergere sulla Camera attiva, attraverso i Gruppi parlamentari, le proposte emendative dei senatori, ha permesso di poterle discutere ed esaminare assieme alle altre. Questa eccezionale collaborazione è legata alla situazione di emergenza. Quindi, non è un dramma per la democrazia; nessun attentato alla Costituzione. Anzi è la dimostrazione che il bicameralismo paritario perfetto è stato fondamentale, perché capace di dare resilienza al Parlamento in questi momenti difficili. Concludo ringraziando il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, di cui sono orgogliosa, perché non si è fatto piegare dalle mille difficoltà incontrate, perché ha lavorato e continua a lavorare senza sosta, unito, al servizio dei cittadini, senza mai perdere l'energia. *(Applausi)*. Quella stessa energia *(Applausi)*. Quella stessa energia con cui siamo entrati il primo giorno in questi palazzi. Un Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, che è stato fondamentale nella risposta decisa e di qualità a questa grave crisi pandemica. Persone che hanno la tenacia e la visione che serve a costruire un Paese sano, forte, moderno da lasciare alle prossime generazioni.

È stato un anno talmente forte che non potremo più tornare a vivere come prima e non potremo nemmeno più economicamente permetterci di pensare che basterà riprendere dal 2019, da dove avevamo interrotto le nostre abitudini.

di chi ha sofferto, di chi sta ancora soffrendo, di chi ha fatto sacrifici e ancora ne sta facendo di enormi, ma soprattutto una scelta necessaria perché se non cambiamo paradigma, se non cambiamo l'approccio ai problemi, rischiamo di far soccombere l'Italia.

se non prendiamo questa situazione molto sul serio, se non affrontiamo i problemi che da molti decenni sono sul tavolo, ma soprattutto se non cominciamo a crescere in maniera decisa, non saremo in grado di sostenere questo enorme debito. Lo diciamo noi, ma lo dicono anche economisti assolutamente illustri e da ascoltare, come Draghi e il governatore

da una giustizia più equa e più veloce al rapporto della pubblica amministrazione con le imprese e con le famiglie, al rapporto dei contribuenti con il fisco e del fisco con i contribuenti. Dobbiamo riformare il lavoro in modo tale che lavorare sia più produttivo e che gli ammortizzatori sociali servano allo scopo di reimmettere le persone nel mondo del lavoro. È necessario, quindi, affrontare tutte le riforme che da anni sono sul tavolo, che da anni l'Europa ci raccomanda, ma per le quali, forse, non abbiamo mai avuto la forza e la stabilità politica neanche il coraggio per dire no quando era necessario. Ricominciare a crescere vuol dire non accontentarsi di ripristinare quella crescita simile alla stagnazione che avevamo fino al 2019 probabilmente nemmeno accontentarsi degli effetti previsti nei documenti del Governo, cioè dell'effetto positivo aggiuntivo sulla crescita che il Piano nazionale di ripresa e resilienza

riusciremo a riportare il rapporto debito PIL nel breve termine a meno 5 punti percentuali e nel medio, sul decennio, ai livelli ante crisi. la vera sfida, che dobbiamo avere assolutamente presente: dobbiamo riassorbire l'enorme divaricazione che abbiamo creato quest'anno con i 108 miliardi di scostamenti, votati anche dalle opposizioni, che hanno portato il *deficit* a meno 10,8

il Governo e il Parlamento dovranno spostare risorse e lavoratori e convertire le competenze verso le nuove economie emergenti. Sarà una scelta comunque faticosa, forse una scelta che avremmo dovuto anticipare nella formazione delle persone che in questa fase erano ferme e che probabilmente erano già disponibili a dedicare del tempo alla loro formazione verso le nuove economie. Lo *shock* ha già provocato la digitalizzazione e la trasformazione dei processi. Una parte sarà determinata dal Next generation EU, ma, inevitabilmente, parte

da molto prima della crisi, insiste sul piano *shock* per l'Italia. Se non investiamo e non mettiamo le aziende, quindi gli investimenti privati e pubblici, nelle condizioni di generare un movimento attivo verso la crescita, non saremo capaci di uscire

pur nella fatica enorme di quest'anno, è stata una scelta semplice, ma la scelta che dobbiamo fare, da gennaio in poi, è molto difficile,

in questa fase, chiedendo in maniera veemente, ma volevamo essere certi di essere pronti ad affrontare questa crisi. Questo perché il dubbio di non essere pronti ci è venuto prima di leggere la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prima di sobbalzare nel letto - vista l'ora - leggendo quell'emendamento che avrebbe voluto sostituire *task force*, Governo e pubblica amministrazione con una *task force* di trecento esterni. Il dubbio ci era venuto già leggendo la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza a ottobre, quando non prevedeva, se non come scenario peggiore, la seconda ondata Dal punto di vista macroeconomico, questo è stato più o meno ripreso nel perimetro, ma dal punto di vista delle misure di contrasto non era stato adeguatamente previsto. La dimostrazione l'abbiamo avuta nel panetto dei quattro decreti-legge ristori e nel ritardo di un mese dell'approdo del disegno di legge di bilancio alla Camera, che ha comportato il fatto che oggi siamo qui a dare la fiducia a ridosso dell'esercizio provvisorio, senza aver potuto discuterla. Il dubbio che ancora non abbiamo esattamente chiara la portata della sfida ci viene anche dalla manovra di bilancio. È pur vero che ci sono degli elementi molto apprezzabili, come l'aver introdotto in unico quadro di finanza pubblica sia le risorse nazionali che quelle europee, ed anche l'aver previsto un *mix* di prestiti - quindi di maggior *deficit* - e di sovvenzioni, ma la composizione della manovra ci lascia alcune perplessità importanti. La prima è l'ammontare delle misure minori introdotte: facendo una somma, sono quasi 8 miliardi di misure minori. Non tutte sono negative, anzi, ma sono sicuramente frammentarie e disomogenee; qui ancora non si vede la linea strategica e i semi della svolta. Molta parte della manovra è dedicata a ripristinare e a proseguire le risorse tampone dei decreti-legge cura Italia, ristori e agosto: quindi la stessa mentalità, la stessa prospettiva di solo aiuto e di sola sovvenzione anche per il futuro. Ma soprattutto ci sono delle criticità sul futuro: anticipiamo con il Fondo di rotazione le risorse del Next generation EU, e lo facciamo impegnando risorse per una riforma fiscale che ancora non c'è,

perché sul Mezzogiorno investiamo 16 miliardi in tre anni per la decontribuzione decidendo di non investire miliardi sul credito d'imposta per gli investimenti, quando tale credito d'imposta avrebbe garantito investimenti reali e per il futuro, mentre il credito di imposta sugli *stock* esistenti non fa altro che consolidare uno *status quo*, senza innescare nessun cambiamento e nessuna prospettiva in tal

Sappiamo anche che le riflessioni possono essere risolte: una infatti l'abbiamo risolta, quella della *task force*. Nella legge di bilancio c'è una cabina di regia incardinata presso la Ragioneria generale dello Stato, che farà monitoraggio e rendicontazione del nostro piano per il futuro. Questo è il modo di procedere.

e di mettervi davanti alle vostre responsabilità. Due anni fa per molto meno il PD ha inscenato anche qui un teatrino, lamentando i pochi spazi messi a loro disposizione, e addirittura è un ricorso alla Corte. sono piene le pagine dei giornali - sono saliti addirittura sul tetto della Camera per protestare contro la ormai invasiva richiesta di fiducia posta su ogni provvedimento. Oggi vi do una notizia: siete arrivati probabilmente a 33 richieste di e quindi credo non vi avanzi tempo neppure di discutere di temi come democrazia, trasparenza, temi che avete messo in secondo piano rispetto al mantenimento del vostro *status* di parlamentari.

ma soprattutto - cari colleghi - cito il balletto per le vostre poltrone. Siete stati impegnati in operazioni tattiche più che strategiche. Peccato che a pagarne il prezzo è questa Nazione di cui noi facciamo orgogliosamente parte e che cerchiamo, proprio nell'interesse collettivo, di migliorare e tenere a galla. Voi invece vi siete lasciati abbindolare

la nostra paura è che, se ne avrete anche 207 del *recovery fund*, li userete con la stessa logica spartitoria, inutile e dispersiva con cui li avete usati. Non farete un gran bene a questa Nazione. Temo che l'emergenza sia non la pandemia che ci ha che ci ha colpiti, ma il fatto che voi non siete in grado di gestirla e quindi la vera fiducia - la citava prima il senatore De Bertoldi - deve essere non quella che chiedete ripetutamente a noi e anche oggi, ma quella che dovreste avere il coraggio di chiedere agli italiani. E allora lì vi accorgereste che forse

se comparati, invece, con le risorse che utilizzate per altro e al fatto che la manovra è di 40 miliardi. Ci sono 2 miliardi per il sostegno di quelle imprese. Signori, noi non siamo come voi, e non lo siamo mai stati. Abbiamo sempre anteposto l'interesse nazionale al nostro interesse particolare: è una cosa che voi non potete dire e non riuscite a spiegare. È per questo che oggi non c'è la diretta televisiva. televisiva. Non è un caso nemmeno che oggi il vostro *leader*, il Presidente del Consiglio, alle ore 11, durante le nostre dichiarazioni di voto, sia impegnato in una diretta televisiva. *(Applausi)*. È un modo per distogliere l'attenzione dalle vostre responsabilità, dal vostro imbarazzo e dall'inettitudine del Governo. L'unico atto serio che potete fare dopo l'approvazione di questa non manovra è rimettere il vostro mandato e fare in modo che siano gli italiani a scegliersi il loro Governo e sicuramente tante delle vostre facce non compariranno più in quest'Aula. Senatore De Carlo, la ringrazio per il perfetto rispetto dei tempi. Lei, d'altronde, è abituato ai *record*: non ricordo altri parlamentari che nella stessa legislatura

intervengo a nome del Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE), di cui mi pregio di essere componente, per confermare la fiducia al Governo e ringraziarlo per aver raccolto numerose istanze che abbiamo posto proprio in nome e per conto degli italiani all'estero. Sono esattamente nove. è stata l'aver ripristinato l'esenzione IMU per i pensionati italiani nel mondo. Anche se solo per il 50 per cento, è un passo in avanti, e noi pensiamo e speriamo di completarlo.

di Ministri e Sottosegretari per i rapporti con il Parlamento, e al ministro Amendola, per avere interloquito con la Commissione europea su questo punto. È molto importante per i nostri pensionati italiani all'estero, che venivano discriminati rispetto ai pensionati in Italia. In secondo luogo, sono state aumentate le risorse destinate agli enti gestori, che sono molto importanti all'estero, perché promuovono l'insegnamento della lingua italiana nel mondo. Allo stesso tempo è stato confermato il fondo per la lingua e la cultura italiana all'estero. È un vanto di questa maggioranza.

Non parlo degli italici di provenienza, ma proprio di cittadini italiani, 6 milioni sono iscritti all'AIRE.

- è l'aspetto che ci interessa direttamente come connazionali all'estero - possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative di utilizzo previste, dello sconto in fattura o della cessione del credito nei casi in cui non abbiano redditi in Italia, al di là di quello fondiario o degli immobili da ristrutturare. Faccio notare che moltissimi italiani all'estero sono proprietari immobiliari in Italia e, quindi, l'estensione a loro del superbonus per le detrazioni è particolarmente benvenuta. Sono state inoltre finalmente confermate le misure per facilitare il rientro in patria dei cervelli, in particolare di coloro che hanno dimostrato, rientrando in Italia, un interesse vero a restare, perché possono dimostrare di avere figli, di possedere abitazioni, di essere intenzionati a rimanere in Italia. Noi abbiamo combattuto questa battaglia accanto ai nostri colleghi alla Camera dei deputati e siamo molto contenti che finalmente siano state recepite le relative istanze. Ulteriori fondi sono stati destinati all'assunzione di nuove risorse umane per la rete consolare: si tratta di circa 150 unità tra impiegati di ruolo e contrattisti; personale che, una volta preso posto nelle varie sedi diplomatico-consolari, servirà a rendere più agile e veloce il lavoro. Si tratta, quindi, di un ulteriore servizio per gli italiani all'estero.

che abbiamo solo noi; i francesi hanno mutuato dagli italiani la rappresentanza istituzionale dei francesi all'estero e hanno previsto una rappresentanza parlamentare al vertice e un Consiglio generale dei francesi all'estero, che è stato copiato dal nostro Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Si sono scordati la parte più importante che noi, da veri democratici, apprezziamo e difendiamo, e cioè i Comites, quelle rappresentanze che, come come i Comuni in Italia, vengono utilizzate in ogni circoscrizione consolare in cui risiedono più di 25.000 italiani - quindi moltissime nel mondo - per rappresentarne gli interessi. I Comites erano bloccati da dieci anni. Nonostante una legge ordinaria che li finanzia e ne prevede a scadenza quinquennale il rinnovo, sono bloccati da dieci anni, ma finalmente nel 2021 gli italiani all'estero potranno rieleggere le loro rappresentanze di base in tutte le circoscrizioni consolari. I Comites sono un esercizio democratico estremamente importante e finalmente con quest'azione potranno essere rinnovati. Da dieci anni era bloccata la Conferenza permanente Stato-Regioni-Provincie autonome-CGIE,

che hanno, attraverso le loro amministrazioni, contatti diretti con le comunità degli italiani all'estero. Questa misura è particolarmente benvenuta. L'ultima - ma non per importanza, almeno dal punto di vista personale - è una battaglia storica che ho portato avanti per dieci anni ringrazio il collega l'onorevole Mario Borghese, anche lui del Movimento associativo italiani all'estero (MAIE), di aver fatto proprio alla Camera dei deputati; soprattutto però ringrazio la maggioranza e questo Governo di averla accolta. Finalmente verrà riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano la ristorazione italiana all'estero: i commi dal 1144 al 1848 definiscono un intervento organico che servirà a a istituzionalizzare, riconoscere, tutelare e promuovere il vero *made in Italy* agroalimentare. Faccio notare che noi siamo fieri delle attività di contrasto all'*italian sounding* che vengono portate avanti all'interno del nostro territorio, ma siamo totalmente inermi rispetto a quello che succede all'estero. Abbiamo fiere mondiali molto importanti in cui i nostri produttori hanno degli *stand* accanto ai quali ci sono *stand* di *italian sounding,* magari anche più consistenti, e non possono fare niente. Finalmente è stato riconosciuto - abbiamo cercato di spiegarlo per dieci anni - che i veri ambasciatori, i veri difensori dell'italianità sono gli italiani all'estero, i ristoratori, i titolari di esercizi di pizzeria, i titolari di esercizi di gelateria;

eccellenze. Si crea finalmente un nuovo canale di distribuzione dei nostri prodotti all'estero, dove siamo deboli nella grande distribuzione organizzata. Si di un canale che era a nostra disposizione e che nessuno aveva mai avuto l'intelligenza di comprendere e valorizzare. Finalmente questo

alla rete diplomatico-consolare per gli aspetti di sua competenza, ma - soprattutto - alla rete delle camere di commercio all'estero. Queste nostre tre reti all'estero, che sono le uniche che abbiamo, finalmente fanno squadra con la rete, che c'era e che nessuno voleva vedere e aveva avuto il buon senso di riconoscere,

Finalmente l'abbiamo anche noi: sarà scritto nella legge, c'è un piccolo bilancio a disposizione per i prossimi tre anni e l'epicentro sarà nazionale della ristorazione italiana nel mondo (stati generali della ristorazione), che si terrà in Italia o all'estero una volta l'anno. Anche per questo, siamo particolarmente contenti di dare la fiducia alla manovra in esame. Vorrei dedicare questa vittoria a un ben più emerito collega che ha calcato questo pavimento per tanti anni, dedicando la sua vita alla causa degli italiani nel mondo, il quale oltre vent'anni fa propose proprio questa misura. Finalmente ci siamo riusciti.

Signor Presidente, il voto dei senatori del Partito Democratico sul disegno di legge di bilancio del 2021 sarà un voto politico di rinnovata fiducia al Governo e insieme di responsabilità, per impedire al Paese l'esercizio provvisorio. Il disegno di legge di bilancio è stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati, mentre il Senato ha concentrato il suo intervento nello spazio ridotto di poche ore. Su questa anomalia dobbiamo saper riflettere con serenità. Non ha senso farne oggetto di propaganda, come le opposizioni sono sempre tentate di fare, ma non sarebbe ragionevole rimuovere un *vulnus* obiettivo che non possiamo, né dobbiamo considerare un momento ordinario della vita delle istituzioni. Approvare la legge di bilancio in un tempo tanto breve, senza alcuna possibilità di porvi mano, è una serie anomalia. Sappiamo tutti in quale rilevante misura il *virus* e la pandemia stanno condizionando l'attività del Parlamento, rendendo possibili procedure singolari che, in altre circostanze, non sarebbero considerate corrette. Ma, come poco fa ci ha ricordato la senatrice Gallicchio, i tempi che hanno contratto l'*iter* di esame del disegno di legge di bilancio sono dovuti alla straordinarietà della crisi sanitaria. sanitaria. La stessa distribuzione dei senatori, divisi tra Aula e tribune, è un fatto che condiziona i nostri dibattiti e conferma plasticamente la straordinarietà della situazione. Sono tutti campanelli d'allarme, avvisi di una lunga malattia delle istituzioni che sarebbe pericoloso trascurare ancora. La gravissima crisi che stiamo vivendo ci dice che l'Italia soffre di punti di debolezza più rilevanti di quelli di Nazioni simili a noi ed egualmente toccate dal virus. Il nostro punto debole più serio è la fragilità dello Stato, la ridotta efficienza della macchina pubblica, l'inadeguatezza del quadro normativo e la debolezza del sistema politico. In cima alla crisi dello Stato c'è il progressivo invecchiamento di un ordinamento che, senza riuscirci, abbiamo più volte cercato di aggiornare alle esigenze dei tempi. Ed è in questa terra di nessuno, tra riforme mai fatte e la pressione degli avvenimenti, che da qualche decennio l'Italia sta procedendo con soluzioni pragmatiche, operando per prassi con modifiche, anche profonde, al suo ordinamento. Cambiare il bicameralismo paritario, rafforzare, in una visione bipolare, la stabilità del Governo e il sistema delle garanzie può aiutare l'Italia a essere più libera, più forte, più prospera; ma ottenere un nuovo equilibrio tra i poteri dello Stato in via di fatto, operando per prassi e non attraverso le procedure costituzionali, espone a rischi consistenti la nostra democrazia perché non sappiamo come questi precedenti potranno essere usati in futuro. *(Applausi)*. Negli ultimi decenni, sia la destra sia la sinistra hanno largamente tollerato la prassi che ha fatto del Governo il primo titolare del potere legislativo. E, sempre per prassi, il Parlamento non è più al centro del nostro ordinamento, ed egualmente per prassi il Presidente del Consiglio non è più *primus inter pares*, ma pian piano è diventato un vero e proprio capo del Governo. Se questo processo è andato tanto avanti, anche il Parlamento ha le sue responsabilità per non essere riuscito a difendere le sue prerogative. Il monocameralismo alternato che stiamo consumando sulla legge di bilancio è la replica di una prassi messa in atto da altri Governi di diverso colore politico, tutti spinti da emergenze che sono sembrate incompatibili con i tempi lunghi del lavoro parlamentare. Tra poco i senatori del Partito Democratico voteranno a favore dell'approvazione della legge di bilancio, e per tutti noi vale il dovere di lealtà nazionale, nel senso che non si possono mandare all'aria i conti dello Stato per un groviglio di carattere formale. Nel lento declino del nostro ordinamento dobbiamo, però, impedire Nel lento declino del nostro ordinamento dobbiamo, però, impedire che quanto legato a un'emergenza grave e di lunga durata venga utilizzato come precedente. La Costituzione vuole che le due Camere partecipino a pari diritto non solo all'approvazione finale degli atti legislativi, ma anche alla loro elaborazione in Commissione e in Aula, e violare questo principio è un *vulnus* che non si può ripetere. Egualmente non possono valere come precedente le eccezionali modalità con le quali è stato approvato il decreto-legge sui cosiddetti ristori. In quel oltre alle note criticità di tutti i maxiemendamenti, sono stati inseriti i contenuti di quattro decreti-legge attraverso la loro trasformazione in emendamenti al testo finale. Non sappiamo come la dottrina e la giurisprudenza classificheranno questa innovazione, ma ogni decreto-legge è un provvedimento a sé stante, che poggia su propri specifici requisiti di necessità e urgenza. Metterli insieme in un'unica legge di conversione è una forzatura ardita, certamente rischiosa per il precedente che può determinare. Le grandi crisi non solo possono provocare l'obiettiva necessità di misure eccezionali, ma, se affrontate con responsabilità, possono stimolare riforme profonde, grandi cambiamenti e nuovi impulsi alla crescita e allo sviluppo. Giorni fa è stato ricordato che il debito pubblico può essere buono, se indirizzato verso spese produttive, ma può essere cattivo, se sprecato alla ricerca del consenso. Uguale sorte può toccare alle riforme modernizzatrici di cui abbiamo un grande bisogno, ma che, come il debito, possono essere riforme buone o meno buone: sono buone le riforme approvate dal Parlamento secondo le regole della Costituzione; sono fragili e rischiose le riforme adottate in via di fatto per prassi, emergenza dopo emergenza, in un piano inclinato di cui è difficile vedere l'esito finale. Per gli italiani questi sono tempi difficili, di grande incertezza e grande preoccupazione per il futuro. Siamo sospesi tra il timore per il virus e l'assenza di informazioni sicure sul lavoro e sull'economia e abbiamo tutti, soprattutto noi parlamentari, ciascuno per la sua parte, il dovere di aiutare l'Italia a capire dove stiamo andando e dove ci sta conducendo l'insieme dei provvedimenti che il Governo e il Parlamento stanno adottando. L'uscita dalla crisi non sarà rapida e il grande lavoro di rilancio non si concluderà nel poco tempo che ci resta in questa legislatura. In prospettiva, i tempi lunghi della crisi sanitaria e delle sue conseguenze economiche e sociali ci impongono di garantire, al di là del succedersi dei Governi e delle legislature, continuità alle linee di fondo dell'azione dello Stato. Per un Paese in difficoltà, come è oggi l'Italia, una delle parole chiave è continuità, continuità delle grandi scelte dello Stato. Un'uscita Un'uscita positiva dalla crisi è quindi nell'interesse, sia della maggioranza che oggi governa, che dell'opposizione che potrebbe governare domani. Insieme dovremo fare tutto quel che possiamo per non sprecare i talenti che ci offre una difficile congiuntura che, oltre al grande dolore per i tanti morti che abbiamo avuto, ci porta anche un'occasione di ripresa e di cambiamento. Sappiamo che all'Italia servono un debito buono e buone riforme. Su questi due obiettivi non dividiamoci e riserviamo la lotta politica ad altro. *(Applausi)*.

Signor Presidente, cari colleghe e colleghi, se rimanessimo fedeli al politicamente corretto dovremmo dire - come hanno fatto sinora molti colleghi - che oggi discutiamo la legge di bilancio. Oggi non stiamo discutendo un bel nulla: siamo chiamati a ratificare decisioni prese altrove, a mettere un sigillo sopra un pacco che non abbiamo nemmeno potuto aprire. la prima forza politica del Paese, in questo ramo del Parlamento oggi viene impedito di dare un contributo attraverso i suoi rappresentanti. È una violazione palese dell'articolo 72 della Costituzione, come ha ricordato poco fa il senatore Zanda, che ringrazio.

denunciò alla Corte costituzionale la compressione dei tempi due anni fa in quest'Aula. La doppia lettura serve non a tutelare le opposizioni, ma a migliorare la qualità della legislazione, anche correggendo eventuali errori. qui di errori ne sono stati fatti tanti, come dimostra il fatto - non ha precedenti - che oggi voi votate una legge di bilancio con il buco: d'altronde, non tutte le ciambelle riescono col buco, anche se il buco non è di qualche decina di migliaia di euro, ma è di 1,5 miliardi. Vi siete dimenticati migliaia di lavoratori dipendenti che guadagnano tra i 28.000 e i 40.000 euro, ai quali avete promesso un *bonus* senza avere prima trovato i soldi. Votate una legge piena di errori, che vi costringe a intervenire nelle ultime ore dell'anno con un nuovo decreto, un decreto tampone: una velocità e un'organizzazione che, purtroppo, non abbiamo visto con i tamponi che servivano nei mesi scorsi per tracciare i contagi. Non siete stati neanche in grado di fare i conti e quindi vi regaleremo un pallottoliere. Più che un percorso legislativo lineare, costruite una *matrioska*, con una legge dentro l'altra ma, quando si arriva all'ultima bambolina, c'è il nulla. Siamo alla trentasettesima fiducia, praticamente ormai ne votiamo una per ogni provvedimento. questa la strategia del Governo: esautorare il Parlamento dei suoi poteri, svuotarlo delle sue prerogative e umiliare le Camere. *(Applausi)*. Questa legge avrebbe dovuto gettare le basi per la ripresa della nostra economia, ma continuate con la politica dei *bonus*. Votate una legge simbolo di una maggioranza politica, che non esiste più. Le vostre divisioni, la vostra ricerca di poltrone, le vostre partite a scacchi, le vostre guerre di potere, le vostre battaglie per la *leadership* tengono in ostaggio gli italiani, già in ginocchio per la pandemia *(Applausi)*. E avete addirittura riportato nel dizionario della seconda Repubblica la parola rimpasto. Non si può essere contemporaneamente di lotta e di Governo, o meglio: non si può essere di lotta e di Governo nell'anno della pandemia, mentre gli italiani muoiono di coronavirus e rischiano di morire di fame. Non si può essere di lotta e di Governo mentre i negozi chiudono e si può essere di lotta e di Governo mentre i negozi chiudono e si creano le file alla Caritas e alle mense dei poveri. *(Applausi)*. È comodo essere al Governo e fare il controcanto ogni giorno, ma chi è al Governo deve dare delle soluzioni, se è in grado di farlo, altrimenti lasci il passo a chi è capace. Anche il *recovery plan* è nel caos e addirittura lo stesso ministro Gualtieri ha ammesso che, continuando così, rischiamo di perdere i soldi del *recovery*. Altro che CIAO: questo *recovery plan* Con una democrazia amputata, tra DPCM e stato di emergenza, con il PIL peggiore d'Europa, con il *deficit* alle stelle e in costante crescita, il Governo Conte prosegue a fare passerelle a favore di telecamera, per i TG serali, e si dimentica del Paese reale. Persino stamattina, mentre discutiamo della legge più importante dell'anno, il Presidente del Consiglio, invece di essere qui, nella casa degli italiani, sta preparando una conferenza stampa per fare il suo *show* di capodanno il totale disprezzo del Parlamento. Quindi lo invitiamo a rinviare alle ore 15 il suo *show*, per venire subito qui, in Parlamento. Avremmo potuto creare un'Italia competitiva e invece avete annaffiato un deserto, creato da chiusure decise contro la logica, seguendo la giungla dei codici Ateco e degli algoritmi. Quando hai il deserto, puoi innaffiarlo quanto vuoi con l'assistenzialismo, ma non crescerà comunque più nulla. Avevate un'occasione storica, poteva essere la stagione del grande riformismo, coinvolgendo innanzitutto i privati, che invece sono completamente assenti, perché per voi il privato è da contrastare a prescindere. *(Applausi)*. Avete finanziato con 4 miliardi di euro la misura fallimentare del reddito di cittadinanza e avete mezzo miliardo di euro per le politiche attive del lavoro. Pensate di gestire il Paese con mance e mancette: questa è la differenza tra noi e voi. Voi pensate di andare avanti regalando caramelle: noi invece vogliamo creare la fabbrica delle caramelle, perché in questo modo si genera ricchezza, si crea occupazione, si reinvestono gli utili, aumenta il PIL ed possibile far decollare il Paese. E se non fosse stato per il centrodestra, avreste preteso il pagamento delle tasse anche da quei lavoratori autonomi e da quelle partite IVA che avete messo in ginocchio e nelle condizioni di non lavorare. L'anno bianco fiscale era il minimo sindacale, ma non è un vostro risultato: è un successo del centrodestra. *(Applausi)*. Muore l'economia, muoiono purtroppo ancora gli italiani. Israele ha vaccinato mezzo milione di persone in dieci giorni in Italia il commissario Arcuri si vanta per gli appena 8.361 vaccini effettuati: un nonnulla. Stamattina leggiamo di un fantomatico piano B: chiamatelo direttamente piano F, come fallimento. *(Applausi)*. E nel disordine più totale, parte della maggioranza ha armato le tastiere dei fanatici, come i no vax, e addirittura una ragazza coraggiosa come Claudia, la prima ad essere vaccinata, invece di essere applaudita e guardata come esempio di coraggio, viene attaccata e minacciata. I vostri errori sono lo specchio della sciatteria: non ve li perdoniamo, perché sono figli dell'arroganza e della superficialità. Alla vostra fiducia effimera in quest'Aula corrisponde la sfiducia degli italiani e non vediamo l'ora che abbiate il coraggio di certificarla. stiamo affrontando l'ennesimo voto di fiducia posto da questo Governo. Non possiamo che criticare le procedure con cui si sta esautorando il potere legislativo del Parlamento: continui decreti-legge e voti di fiducia sono ormai la regola. A queste procedure straordinarie si sono aggiunti i DPCM del presidente Conte, spesso ingiustificati e inopportuni. La manovra è stata portata all'attenzione della Camera dei deputati con trentacinque giorni di ritardo - come hanno ricordato molti colleghi - e al Senato il 28 dicembre. Il vice ministro Misiani ha confermato che la legge di bilancio che stiamo per ratificare è sbagliata e andrà corretta. Queste procedure, questi abusi, queste inefficienze sono già sufficienti per poter esprimere un giudizio negativo sull'operato di questo Governo. Ciò che ci preoccupa di più, però, non è il metodo con cui governate, ma sono i contenuti dei vostri provvedimenti. Non ci piace e non ci convince come avete affrontato l'emergenza sanitaria nel nostro Paese. Non ci piace e non ci convince come avete affrontato la riapertura delle scuole a settembre. Non ci piace e non ci convince come avete affrontato la gestione del trasporto pubblico locale. Non ci piace e non ci convince come avete gestito i decreti ristori. E, soprattutto, Presidente, non ci piace non ci convince la politica economica di questo Governo. Ma veramente pensate che con i bonus, i sussidi, il reddito di cittadinanza e di emergenza, con il *click-day* e con il *cashback* riuscirete a risollevare le sorti della nostra economia? Riuscirete a salvare il lavoro di centinaia di migliaia di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi? Siete veramente così sprovveduti e lontani dalla realtà? Girate le nostre strade, parlate con i cittadini e confrontatevi con le categorie; la situazione economica è drammatica e quella sociale è esplosiva. Il Parlamento ha autorizzato manovre a debito di oltre 100 miliardi in pochi mesi. Voi state gestendo male, malissimo questa opportunità; la state sprecando, perché la vostra mentalità di fondo è sbagliata. Il MoVimento 5 Stelle vive nel suo mondo di decrescita felice e di intero popolo che dovrebbe vivere di sussidi e reddito di cittadinanza: una follia che economicamente non regge e che ci porterebbe al disastro. Il PD e LeU portano avanti la solita teoria della raccolta insostenibile delle tasse per poi operare una redistribuzione del reddito con i bonus. Ma voi non redistribuite ricchezza: redistribuite povertà e miseria. La montagna di ulteriore debito pubblico che il Parlamento ha autorizzato doveva essere indirizzata non a bonus e sussidi, ma alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle attività che a fatica cercano di sopravvivere. Il denaro speso meglio da uno Stato efficiente è quello lasciato nelle tasche dei cittadini. Deve circolare liberamente. È una follia sottrarlo ai cittadini con mille adempimenti fiscali per poi redistribuirlo con i bonus. Questo modello non regge: è stupido, inefficace e produce adempimenti burocratici complessi e costosi. Voi state seppellendo il Paese sotto una montagna di debito pubblico, gettando al vento decine e decine di miliardi. Le vostre misure non sono efficaci e lo dimostrano i dati: il turismo è in ginocchio, le attività commerciali chiudono i battenti a migliaia, gli autonomi non possono lavorare. Noi vogliamo che queste attività sopravvivano e l'unico modo è esentarle dal pagamento di tasse che non sono in grado di pagare. E non possono pagarle non perché sono dei farabutti o degli evasori, come li amate dipingere voi della sinistra, ma perché lo Stato (il Governo) ha chiuso le loro attività. State molto attenti, perché sono loro che mantengono in piedi le casse dello Stato. Più attività farete fallire, minore sarà anche il gettito, minori saranno le risorse a disposizione dello Stato per finanziare stipendi pubblici e servizi ai cittadini, maggiori saranno i crediti deteriorati e le risorse che dovrete stanziare per risanare le banche; state giocando col fuoco. Cosa accadrà poi quando sbloccherete i licenziamenti? Prima o poi ci arriveremo a quella data. Cosa accadrà quando non avrete più possibilità di finanziare la cassa integrazione, perché non avrete più risorse? Cosa farete quando padri di famiglia non avranno più un reddito, un'attività, un lavoro per pagare l'affitto e mantenere la propria famiglia? Cosa farete quando decine di migliaia di cartelle esattoriali pioveranno sulle teste dei cittadini? Le state solo rinviando e la montagna aumenta. Cosa farete quando a Bruxelles vi diranno che non potremo più fare altro debito e vi chiederanno di restituire quanto vi è stato concesso? Quella data prima o poi arriverà. I decreti ristori e questa manovra di bilancio, infarciti di centinaia di misure microsettoriali e localistiche, sono una vera e propria vergogna. Lo sono soprattutto in questa fase drammatica che stiamo vivendo. Ogni singolo centesimo andava utilizzato con grande oculatezza e rispetto nei confronti degli italiani. Non lo avete fatto e non so se ve ne pentirete, ma sicuramente tutto il Paese ne pagherà le conseguenze. Abbiamo insistito perché i decreti ristori non si basassero sui codici Ateco, ma sul calo di fatturato di tutte le categorie di autonomi. Non ci avete ascoltato; avete dato miserie a pochi e nulla alla maggior parte delle categorie. Abbiamo cercato su ogni provvedimento di offrirvi la nostra collaborazione; non ci avete quasi mai ascoltato. Siamo però orgogliosi di aver ottenuto l'esonero totale nel 2021 dei contributi fissi per autonomi e professionisti che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 33 per cento e abbiano avuto un reddito non superiore a 50.000 euro euro (emendamento Garavaglia alla legge di bilancio). *(Applausi)*. Siamo orgogliosi di aver cancellato l'obbligo della partita IVA per il volontariato (emendamento Garavaglia alla legge di bilancio). Siamo orgogliosi di aver ottenuto l'abbattimento degli oneri di sistema nelle utenze elettriche di tipo commerciale per le attività che non hanno potuto lavorare (emendamento Arrigoni, Romeo e del centrodestra al decreto ristori). Siamo orgogliosi di tutti quegli emendamenti che miravano alla riduzione della pressione fiscale, ma siamo consapevoli che molto di più andava fatto. Molto di più è necessario al nostro sistema economico e produttivo per risollevarsi. Voi non vi state dimostrando all'altezza di questo compito; noi abbiamo il dovere di continuare a insistere perché cambiate rotta, abbiamo il dovere di farci trovare pronti quando toccherà a noi la responsabilità di governare. E lo saremo. Speriamo solo di non arrivarci troppo tardi, quando di questo Paese e della nostra economia rimarranno solo macerie. Questa legge di bilancio rappresenta l'ennesima occasione persa; non è adeguata ai drammatici momenti che stiamo vivendo. Il nostro Paese merita di meglio e questo Governo non merita la nostra fiducia. *(Applausi)*.

colui che mi ha preceduto ha detto un sacco di inesattezze; cercherò di argomentare puntualmente sul suo intervento. Il decreto rilancio, il decreto liquidità, il decreto agosto, il decreto ristori...

gli imprenditori italiani sono stati aiutati a superare questo lungo momento di difficile crisi. Devo dire che tra questi quattro provvedimenti che ho citato e la legge di bilancio c'è una differenza sostanziale. Con questo testo che stiamo per votare cominciamo a delineare lo sviluppo futuro delle aziende italiane. Sicuramente, è importante il supporto economico statale durante la crisi per evitare il più possibile le difficoltà, ma è anche necessario lavorare con un'ottica di medio-lungo periodo e di questo parliamo oggi. Tutte le norme presenti in questo testo, che si riferiscono appunto alle aziende, sono pensate per l'industria italiana del futuro. Non troverete mai, in un provvedimento di questo Governo, qualcosa che non abbia comunque uno sguardo, anche solo in parte, verso la pianificazione del tessuto industriale di domani. Quando parlo di tessuto industriale, non mi riferisco solamente agli imprenditori e alle loro aziende; qui parliamo di lavoratori, di nuove professioni, di incentivi ad un'industria più verde e tecnologicamente avanzata. Una volta si utilizzava il detto "mettere la chiesa al centro del villaggio". Oggi noi mettiamo l'impresa al centro del sistema Paese. Questo lo facciamo con riforme incisive, che permetteranno all'industria di trasformarsi per saper rispondere alle esigenze dei prossimi decenni. Abbiamo introdotto crediti d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali nel lavoro agile, incentivi per ricerca e sviluppo, per innovazione tecnologica, per investimenti nella *green energy*, nel digitale nonché nel *design*. Tutti i crediti di imposta che verranno maturati saranno duraturi. Sono validi per due anni abbondanti, fino al giugno 2022. Contemporaneamente a questo, manteniamo una potenza di fuoco estremamente elevata per garantire la liquidità delle imprese italiane, prorogando fino a giugno 2021 la garanzia pubblica del fondo PMI su prestiti alle imprese. Questa proroga si aggiunge agli oltre 100 miliardi già prestati fino ad oggi. Non voglio dilungarmi troppo, perché le norme sono veramente tante e articolate, coprendo innumerevoli necessità delle imprese italiane, ma voglio sottolineare come sia stato esteso ancora una volta il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione. Se da una parte, infatti, supportiamo il rilancio aziendale non vogliamo però che nessuno rimanga indietro lasciando a casa i propri lavoratori. Lasciatemi citare un'altra norma presente in questo testo, su cui lavoro da mesi e che ho presentato anch'io personalmente, più volte, a partire dal decreto rilancio. L'Italia ha una grande risorsa, che è l'acqua. Quante volte abbiamo letto o ascoltato che l'acqua è vita. L'Italia è un Paese verde e rigoglioso, cosa che fa dell'acqua una delle risorse principali anche per le energie rinnovabili, tanto che gran parte dell'energia viene prodotta da grandi centrali idroelettriche. però, che certa stampa, di fronte a delle norme più innovative e - devo dire - attese da ormai troppo tempo, si divida per cercare di schernire, come spesso fa, il lavoro del Governo. In questo provvedimento è stato inserito un emendamento alla Camera, che introduce una detrazione di imposta per chi installa vasi da bagno e rubinetteria, proprio per andare incontro alla necessità del risparmio idrico. Ecco, quella che voglio sottolineare oggi è la faziosità di una lettura politica di questa norma, che va travisare quella che è la sua reale finalità. Non toccate questa norma. L'Italia è uno dei Paesi dove si investe di più per il potenziamento della rete idrica a causa dei suoi problemi di dispersione. Secondo i dati Istat, il 37 per cento circa dell'acqua immessa nella rete viene dispersa. In alcune province italiane, si arriva addirittura al 60 per cento. In aggiunta a questo, gli italiani, con il proprio atteggiamento quotidiano nell'uso dell'acqua domestica, contribuiscono a disperdere ulteriormente preziose risorse idriche. Per questo credo che una norma che incentivi l'acquisto di rubinetterie che faranno risparmiare anche il 50 per cento dell'acqua domestica, che altrimenti andrebbe dispersa, siano i benvenuti. Mi direte che 20 milioni per finanziare questa norma sono pochi; intanto, è fondamentale averla inserita per la sua bontà intrinseca. Ovviamente lavoreremo per incrementare i fondi e far sì che migliaia di italiani possano ridurre i propri sprechi. Risparmiare acqua e ritrovarsi con sanitari e rubinetterie di ultima generazione non mi pare una situazione sulla quale ironizzare. È poco? Intanto, partiamo. Concludo, colleghi, auspicando che tutti ci si renda conto degli impegni che il Paese deve affrontare e che ci si cali nei panni del cittadino in difficoltà senza manie di protagonismo e distinguo che non hanno ragione di esistere. Pensiamo ai cittadini, ci hanno mandato qua per questo.

anche questa volta devo cominciare ricordando che un ramo del Parlamento si trova nell'umiliante situazione e condizione di dover approvare un testo su cui non è potuto intervenire minimamente. Questa prassi del bicameralismo zoppo era presente anche prima dell'emergenza sanitaria; basta andare con la memoria alle ultime due leggi di bilancio. Il fatto però che tutte le forze politiche, una volta al governo, usino certe modalità, non è una buona giustificazione e non lo sarà fino a quando non verrà cambiata la Costituzione. Fino a quel giorno vigerà un sistema basato su due Camere che hanno uguali funzioni e prerogative e ogni forzatura in tal senso è una forzatura rispetto al corretto funzionamento democratico. Fatta questa premessa, Presidente, il testo che abbiamo letto va inscritto nel percorso cominciato a marzo per fronteggiare l'emergenza economica. Altri 40 miliardi di euro nel circuito produttivo e per le famiglie, cui, come sappiamo, seguirà presto un ulteriore scostamento di bilancio per indennizzare le categorie che soffrono per via delle restrizioni e delle limitazioni. Il mio Il mio pensiero va qui allo sci e alla montagna, su cui proprio in questi giorni si sta discutendo di quello che succederà dopo il 7 gennaio. Agli interlocutori istituzionali (CTS) chiediamo soprattutto una cosa: risposte certe e in tempi brevi, non come l'ultima volta, che quando le Regioni hanno dovuto attendere quasi un mese per ottenere risposte dal CTS. La montagna richiede programmazione e non si possono cambiare le carte in tavola sempre all'ultimo minuto. Lo sci e il turismo invernale della montagna non sono solo svago, ma un'industria con una filiera molto profonda che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ed è incredibile che questa industria non venga considerata dal Governo. Purtroppo, al momento, io vedo al riguardo solo incertezze; incertezze sulle aperture e sui ristori. colleghi del Parlamento e del Governo, è proprio inaccettabile. Tornando al provvedimento, la sensazione è che manchi un tema forte, un investimento

caratterizzato da uno spezzettamento delle risorse per finanziare una mole forse eccessiva di interventi. È ovvio poi che davanti a un numero così corposo di interventi se ne trovino di positivi, anche se resta più di un dubbio sull'efficacia e sull'impianto della legge. Mi riferisco in particolare alle misure per i lavoratori autonomi, la categoria forse meno raggiunta dallo sforzo di questi mesi, con i primi ammortizzatori sociali e la prospettiva di un anno senza incombenze fiscali per chi avrà segnato importanti cali di fatturato. Bene anche il rafforzamento del superbonus del 110 per cento a condizione che si rifletta anche sulle modalità di accesso perché l'impegno burocratico per attingere a questo beneficio fiscale è davvero molto gravoso, come denunciano praticamente tutti gli operatori del settore. anche tutto il pacchetto di misure volto a rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie, dalla conferma del taglio del cuneo fiscale all'assegno natalità, così come le agevolazioni tributarie per le assunzioni. In questa legge ci sono anche delle misure che interessano da vicino le autonomie e la mia Provincia autonoma di Bolzano. Mi riferisco alla norma sui requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio provinciale, che - è bene ricordarlo - nasce per adeguare l'Italia alle direttive europee, e consentirà alla nostra Provincia di fronteggiare con maggiore efficacia la cronica carenza di personale. Penso anche alle risorse destinate allo sviluppo delle opere legate alle Olimpiadi invernali del 2026, così come alla norma di attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra Governo, Regioni a con la riduzione di 100 milioni di euro del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, a titolo di compensazione per la perdita di gettito a causa dell'emergenza pandemica. È un piccolo segnale che il Governo dà alle autonomie, ma servono ancora sforzi molto più sostanziosi. Su questi punti, in particolare sulla norma delle professioni mediche, teniamo a ringraziare il Governo e la maggioranza per l'attenzione dimostrata. Il compromesso raggiunto è la riprova di un buon dialogo, che speriamo continui anche su altri temi, a cominciare da un maggiore impegno finanziario nel *recovery plan* per la montagna. In conclusione, ci lasciamo alle spalle un anno difficilissimo in cui il Governo ha fatto uno sforzo importante. Tuttavia, nel 2021 quello sforzo rischia di non bastare. Occorre rafforzare gli strumenti per quei settori dove la mortalità delle imprese può essere devastante, come ha ricordato Confesercenti con il suo ultimo studio. Occorre ripensare velocemente il rapporto col fisco e quindi andare avanti con l'impegno per un anno bianco per le partite IVA o per un nuovo saldo e stralcio per chiudere le situazioni sospese. Occorre migliorare la catena decisionale sulle riaperture e sulle restrizioni, perché i tempi, non solo in montagna, sono un elemento essenziale. In ultimo, ma non per ultimo, bisogna fare in fretta e fare bene sul *recovery fund*, su cui si gioca il destino del Paese, delle future generazioni, ma anche il futuro dell'Europa: se l'Italia fallirà, sarà un formidabile argomento per i rigoristi e per coloro che sono contro un'Europa unita. Insomma, nel 2021 facciamo ancora di più, e soprattutto facciamolo meglio.

onorevoli colleghi, il 2020 ci consegna un quadro internazionale nel quale possiamo riconoscere due vincitori e due vinti. Ha vinto la scienza: grazie, scienza. se non vi fosse stato un gigantesco investimento nella farmaceutica, nella sanità e nella medicina, noi oggi saremmo ancora senza una prospettiva di speranza contro il coronavirus. Ovviamente, la strada è ancora lunga, ma il fatto che ci sia un vaccino in un tempo record è un fatto storico. Mi piace pensare che nella corsa al vaccino fatta in tutto il mondo siano arrivati primi - non perché fosse una competizione, ma perché comunque era una sfida epocale - dei coniugi turchi stabiliti in Germania: Ugur e Ozlem, questi i nomi di battesimo. È la storia di un grande Paese che accoglie un'immigrazione di qualità e che ne fa strumento di competitività. La stessa cosa era accaduta nella Silicon Valley. Per me, la stessa cosa dovrà accadere nei prossimi dieci anni in Italia: per questo insistiamo su alcuni provvedimenti da inserire nel Next generation EU. C'è bisogno di fare di questo Paese il luogo del capitale umano, come ha fatto la Germania che oggi ha il quintuplo dei vaccinati dell'Italia. C'è bisogno di scommettere su forme nuove di rapporto tra scienza, ricerca, cultura, capitale umano ed educazione: questo è il punto di partenza del Next generation EU, non una paginetta giustizialista sulla giustizia. Dall'altro lato, grazie Europa. Non si sentono più - in quest'Aula, almeno - i No-vax, eppure si sentivano; e non è più forte come prima la retorica sovranista. Perché? Perché la retorica sovranista si basava su un'inerzia dell'Europa, che c'è stata oggettivamente negli anni passati, e che oggi non c'è stata, perché l'Europa ha messo una incredibile mole di risorse, che va oltre le nostre migliori aspettative: Next generation EU, European Central Bank (ECB), il programma SURE, il MES (con 36 miliardi di euro sulla sanità che potrebbero cambiare la storia della sanità del nostro Paese) e naturalmente la programmazione tradizionale. Ora, la questione è che dobbiamo spendere bene questi soldi, con riguardo a due aspetti: il primo è quello relativo relativo alla visione del Paese. Sulle forme della democrazia, signor Presidente - lo ha riconosciuto anche lei e la ringrazio di questo - oggi abbiamo ascoltato parole per me definitive di un collega, con il quale non sono mancati elementi di divergenza, che risponde al nome del senatore Luigi Zanda. Chi non era in Aula, per cortesia, legga l'intervento del senatore Zanda. Chi non crede a ciò che diciamo noi da mesi, perché siamo quelli che vengono etichettati come irresponsabili e Pierini, non ascolti noi, ma ascolti il senatore Zanda. Dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità delle istituzioni che, al momento, rischia di essere messa a dura prova. *(Applausi)*. Se il Governo giallo-verde fa la legge di bilancio in quarantotto ore al Senato, si va alla Corte costituzionale, come hanno fatto i colleghi del PD nel 2018. Se lo fa il Governo giallo-rosso si sta zitti? Non è possibile. C'è bisogno di un rispetto delle regole indipendentemente da chi afferma per prassi un principio che pure io condividerei, perché se c'è uno in quest'Aula che è a favore del superamento del bicameralismo sono io, ma siccome non ci è riuscito, ahimè, siccome non ci è riuscito, ahimè, oggi il bicameralismo dobbiamo rispettarlo, perché se passa il principio che le riforme costituzionali non servono e basta una prassi, noi stiamo distruggendo questa Assemblea, stiamo distruggendo la nostra credibilità, noi e voi insieme.

dai Servizi segreti, fino alle questioni legate al modo in cui si fa una legge di bilancio. *(Applausi)*. Non è di noi che stiamo parlando, ma della nostra credibilità e della vostra credibilità. canto, bisogna accelerare. Leggo oggi le parole del Ministro dell'economia, che alle 14 riceverà una delegazione di Italia Viva, che non è qui con noi ma sicuramente ci seguirà da casa. è bellissima l'idea dell'accelerazione. Chi come lei, più di me, ama il futurismo sa che l'accelerazione e la velocità sono un mito straordinario. Io sono uno di quelli che hanno chiesto commissari, che hanno chiesto di sbloccare le opere, figuriamoci se sono contrario all'accelerazione. Il 22 luglio in quest'Aula ho chiesto di fare una sessione ad agosto sul Next generation EU, oggi scopro che siamo in ritardo e bisogna correre. Bene. Sul correre siamo tutti d'accordo, ma la mia domanda Perché se si corre nella direzione opposta a quella corretta, per tornare indietro ci vuole il doppio del tempo. La domanda da porsi è se questo debito, buono o cattivo a seconda delle scelte che facciamo - parole con il *copyright* di Mario Draghi - vogliamo affrontarlo o no? Resti agli atti, Presidente, che questa finestra temporale che si apre non è una finestra casuale, è una finestra che per trent'anni non c'è stata. Nessuno ha potuto spendere questi soldi, è chiaro? Ci sono sindaci in tutti gli schieramenti, di destra e di sinistra, ci sono Presidenti di Regione, ci sono amministratori locali: noi non abbiamo avuto mai la possibilità di spendere questi soldi, eravamo bloccati dal Patto di stabilità, dai blocchi lo sappiamo tutti - di destra e di sinistra. Per i prossimi trent'anni non ci sarà possibilità di spendere questi soldi. La finestra temporale è ora ora o mai più, perché poi a un certo punto le porte dell'Europa si chiuderanno. Se siamo in condizione di metterci d'accordo sul fatto che si devono spendere questi soldi sulla cultura, sulle infrastrutture, sull'ambiente, sulle opportunità, siamo credibili, se invece affermiamo il principio che un Gruppo parlamentare, una forza politica non può chiedere conto di come si spendono questi soldi, perché altrimenti disturba il manovratore, stiamo trasformando il Parlamento in un luogo da schiacciatasti, ma - attenzione - non stiamo dando stabilità. Lasciatemelo dire ai colleghi della maggioranza. A chi ci viene a dire che siamo irresponsabili perché mettiamo in discussione la stabilità

Ma c'è una differenza epocale tra la stabilità e l'immobilismo. Una legislatura sta in piedi come una bicicletta: l'equilibrio lo trova se si muove, se riesce ad avere una visione e un orizzonte. Se ci mettiamo in uno stallo, l'immobilismo è esattamente ciò che fa terminare in anticipo la vita di una legislatura.

Oggi sono patrimonio condiviso perché tutte le forze politiche stanno mandando avanti i propri progetti. Venti giorni fa siamo stati etichettati come irresponsabili; stavamo soltanto dicendo la verità. Un grande statista di questo Paese nelle ore più difficili della sua vita

Erano le parole di Aldo Moro nel momento più difficile della sua esistenza, ma sono le parole che dovrebbero ispirare tutti noi. *(Applausi)*. Sono le parole che consegniamo al Governo nell'ultimo intervento di questo 2020 che ci ha visto dire sì convintamente per lealtà istituzionale. Diremo sì anche oggi, ma assegniamo al Governo la responsabilità di decidere cosa fare da grandi, perché siamo stati *partner* di questo passaggio complicato; siamo pronti a lavorare insieme se c'è una visione e un orizzonte sulla base delle cose che abbiamo detto, dell'idea dell'Italia tra trent'anni, di un percorso che ci permetta di spendere bene i soldi, di avere quel debito buono di Draghi. Non saremo mai complici del più grande spreco di denaro che potremo avere nella storia repubblicana. *(Applausi)*. Se vogliamo andare avanti, si va avanti su un progetto. La palla passa al Governo e non più a noi perché noi abbiamo soltanto detto la verità.

la manovra arriva in Aula senza relatore. Su questo vorrei fare una prima riflessione perché non più tardi di un mese fa

addirittura senza aver avuto la possibilità di discutere in Commissione della manovra di bilancio - che, voglio ricordarlo, è l'atto più importante di una legislatura - e addirittura senza avere un relatore in Aula che potesse darci delle indicazioni sul tema della manovra di bilancio. Allo stesso modo, voglio dire anche al presidente della Commissione bilancio di finirla con questi sermoni che ogni volta ci fa prima di venire in Aula dicendo che questa sarà l'ultima volta che ci sarà questo tipo di problema, questo tipo di corto circuito nelle Aule parlamentari.

come accade costantemente in questo ultimo anno, a questa prassi consolidata per cui una sola Camera viene messa nella condizione di lavorare sui provvedimenti, mentre l'altra, come in questo caso oggi il Senato, viene esclusa da qualsiasi decisione, perché non è praticamente a conoscenza di nulla. Su questo Fratelli d'Italia continua ad appellarsi

mentre dall'altra parte il Governo è in altre faccende affaccendato, cioè il teatrino politico che vede contrapposti il *premier* Conte e l'ex *premier* Renzi, che non si trovano d'accordo su nulla. Come abbiamo sentito qualche minuto fa quando prima di me è intervenuto il senatore Renzi, non si trovano d'accordo su nulla, tranne

vale a dire i 209 miliardi che devono interessare il popolo italiano. Invece è in atto una sorta di spartizione di queste risorse e di poltrone su cui ancora non trovate nessun tipo di quadra. Questo lo sta dimostrando un vostro alleato: lo ha detto poco fa in parole povere il vostro Renzi, che grida effettivamente più di qualsiasi altro *leader* di questa maggioranza, ma che è anche il più insignificante di ognuno di voi, perché - come si dice - abbaia alla luna, perché mai e poi mai potrà far cadere questo Governo

e ci troviamo di fronte a degli eventi che sono epocali. Mi riferisco in particolare al fatto che siamo ormai prossimi ad una delle più grandi campagne di vaccinazione della storia repubblicana, all'interno probabilmente probabilmente della più importante crisi economica dal Dopoguerra ad oggi. Invece, in un momento come questo, assistiamo ad uno spettacolo di guerra di potere, a una spartizione di poltrone all'interno di questa compagine di Governo.

che hanno una stella polare, quella dell'assistenzialismo spinto unito ai *bonus,* di cui effettivamente pochi sentivano il bisogno. Ho sentito parlare del *bonus* rubinetti, in un momento drammatico della vita del Paese, del *bonus* occhiali, del bonus *smartphone;* sono misure che in un altro commento storico avremmo anche potuto accettare, ma in questo momento penso che agli italiani interessi più il proprio posto di lavoro. Io penso che gli italiani in questo momento interessi più il rilancio economico e produttivo del sistema Paese per far sì che l'economia possa davvero ricrescere, rinascere, ripartire, per dare una speranza di futuro ai nostri giovani. Non possiamo accettare questa manovra, perché continuiamo a finanziare una misura che è la più assistenziale che possa esistere, cioè il reddito di cittadinanza. Lo scorso anno impegnammo per finanziare questa misura oltre 7 miliardi di euro; quest'anno continuiamo a impegnare oltre 4 miliardi di euro. euro. Un Governo serio si sarebbe messo una mano sulla coscienza e avrebbe preso atto dell'insuccesso della misura. Voi, invece, imperterriti, continuate a fare finta di nulla, pagando con risorse pubbliche gli spacciatori, i mafiosi e persino gli assassini.

Voi non sapete programmare l'oggi, né il domani né il dopodomani. Caro ministro Gualtieri, invece di salutare, ascolti gli interventi che facciamo. Le voglio ricordare che dopodomani, quindi tra due giorni, sono pronti 31 milioni di cartelle esattoriali. Abbiamo detto a più voce e in tutte le lingue di bloccare la partenza di queste cartelle esattoriali, ma dal Governo non abbiamo avuto alcuna risposta. Pertanto, l'auspicio è che lei,

per cento, anche se si poteva fare molto di più, perché serve più tempo per dare respiro all'economia nazionale. Non basta quest'ulteriore differimento al 31 dicembre

Li avete sperperati e continuate a farlo, come dimostrano le ulteriori mance e *bonus* che continuate a dare anche con questa manovra di bilancio.

nella realtà quotidiana. Noi chiaramente non abbiamo mai nascosto la gravità del momento che stiamo vivendo, ma, al contempo,

non è mai di una sola parte politica o di una sola maggioranza, piuttosto che dell'opposizione. Il futuro è di tutti e solo chi sa costruirlo con tutto il popolo italiano rimarrà impresso nella storia della Nazione. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma non saremo mai complici dei vostri disastri. Per darvi la nostra fiducia avremmo avuto bisogno di comprendere la vostra

la straordinarietà del processo di approvazione di questo bilancio è evidente a tutti ed è di per sé un problema oggettivo. Non possiamo, però, dimenticare la pandemia, la situazione del tutto straordinaria in cui ci siamo mossi: almeno quattro manovre in un anno.

Non dico questo per negare il problema che abbiamo di fronte; dico, però - e

Ragazzi, onestà intellettuale per onestà intellettuale. Non volevo polemizzare su questo; volevo, invece, fare un altro ragionamento. C'è un problema che riguarda la qualità della democrazia e il funzionamento delle istituzioni;

ci pone problemi profondamente nuovi: rapporto politica-scienza; rapporto decisione, tempi e funzionamento delle istituzioni. È un tema su cui dobbiamo lavorare e nessuno può scagliare la prima pietra. Mi auguro che si costruisca un percorso per riuscire a dare risposte innovative.

la riforma fondamentale per introdurre equità e giustizia. Una riforma che non possiamo più rinviare e che può rappresentare una vera e propria svolta. Ancora, la proroga del superbonus, ma anche le azioni sul lavoro. Ancora parliamo di assistenzialismo quando cerchiamo una strada per tutelare il lavoro? Non c'è solo la cassa integrazione. Per la prima volta è stata introdotta una forma di cassa integrazione per gli autonomi, e peraltro lo abbiamo fatto insieme, maggioranza e opposizione. Perché

ristori, contributi alle imprese e riduzione del carico fiscale, per dare una risposta strategica e uscire dalla morsa totalmente inadeguata degli Ateco. Ci sono scelte importanti sulla cultura e sulla scuola. C'è il fondo per il programma Next generation EU,

benissimo Industria 4.0 e le ulteriori risorse per Industria 4.0, ma vogliamo decidere qual è la politica industriale e la strategia? Vogliamo investire sulle scienze della vita, sulle biotecnologie, sulle nanotecnologie oppure facciamo una politica a ombrello? Non è statalismo questo, non è statalismo darsi degli obiettivi strategici per fare un salto di qualità nel nostro sistema economico e produttivo in filiere e in modo integrato. È un tema fondamentale per affrontare la trasformazione. Il nostro problema sull'utilizzo delle risorse per me è prima di tutto questo: dobbiamo assolutamente essere in grado di cambiare l'assetto del sistema economico-produttivo del Paese tutte le risorse che investiamo vanno destinate alla trasformazione ecologica e al cambiamento del modello di sviluppo. Questa è la nostra sfida; non abbiamo bisogno di centinaia di progetti. Abbiamo bisogno di concentrare le risorse su questioni strategiche e decisive, che provo a indicare. del Mezzogiorno, non già in chiave assistenzialistica, ma, volendo parlare di turismo, per investire strategicamente su una nuova filiera produttiva ed economica qual è il turismo in un territorio che ha risorse naturali straordinarie. Ma allora bisogna pensare a una piattaforma per il turismo affinché l'*incoming* non lo facciano le piattaforme straniere. Non abbiamo bisogno di investire 200 milioni di euro per fare

non abbiamo camere e alberghi di qualità, né abbiamo reti capaci di aggredire il mercato internazionale. È su questo che dobbiamo investire,

non i tecnici, non riusciremo mai a spendere le risorse, se non attrezzeremo in forme straordinarie la pubblica amministrazione. Questo vale per il centro e vale per i Comuni e per le Regioni. Non abbiamo più persone in grado di fare i piani strutturali per l'urbanistica, è questo il problema; non abbiamo persone che sappiano fare le gare o la direzione dei lavori. Si tratta di un impegno straordinario.

di partiti e non si misura sulle limature tra la mia proposta, la tua proposta e un'altra proposta.

Siamo intervenuti sui farmaci, per ridurre e cambiare il rapporto tra farmaci territoriali e farmaci ospedalieri

farmaci equivalenti dieci volte il loro valore. Dobbiamo togliere i vincoli alle assunzioni di personale, dobbiamo fare una riforma, dobbiamo cambiare.

indispensabile per la tenuta sociale del nostro Paese, necessaria per sostenere misure utili alle famiglie e alle imprese per attraversare questa crisi pandemica.

ha l'impostazione politica e culturale di una coalizione che - non lo dobbiamo dimenticare - si assume la responsabilità di portare l'Italia fuori dalla crisi.

un ruolo fondamentale e decisivo della scienza e della ricerca, che ci mettono oggi nelle condizioni di vedere una luce in fondo al tunnel - ovvero il piano nazionale di vaccinazione, così importante per affrontare questa sfida

una pericolosa iniziativa rigorista, che ci aveva preceduto, in un nuovo volto europeista, in grado di consentire al nostro Paese di attraversare questa crisi. Questi sono due elementi fondamentali. Ricordo l'inizio di questa legislatura, quando qui si applaudiva ad un'azione contro l'Europa che in molti casi rivendicava un ruolo innaturale e disumano delle condizioni di legalità e di sicurezza del nostro Paese.

europeismo e ad una nuova capacità della scienza di farci uscire dal tunnel della pandemia e il Partito Democratico riconosce il lavoro e il contributo che questa maggioranza e questo Governo hanno offerto per portare l'Italia fuori da questa crisi. Dobbiamo abituarci insieme, se vogliamo restituire dignità alla parola politica, ad inquadrare la fase politica che stiamo attraversando, questa è una fase politica inedita per il mondo e per l'Europa. Sarei molto cauto nell'indicare graduatorie, limiti, priorità

la cautela di attendere l'uscita dalla pandemia. Avremo tutto il tempo e il modo per valutare i tassi di mortalità e i limiti delle nostre azioni che riconosciamo, perché dentro una pandemia ci sono limiti evidenti di tutti i governi in Europa. Tuttavia, dobbiamo inquadrare questa fase politica; lo dico nel pieno rispetto delle prerogative delle opposizioni. Sapete che non è questo il punto; ho pieno rispetto delle prerogative delle opposizioni, accettabili lezioni di democrazia o, peggio ancora, confronti tra annualità diverse, perché paragonare la legge di bilancio del 2018 alla legge di bilancio del 2020 è fuorviante e strumentale. È un rigurgito di sovranismo, già sconfitto sia nella dimensione europea che in quella nazionale. *(Applausi)*. Se noi siamo qui oggi, se il Governo e la maggioranza hanno introdotto azioni complesse e difficili per tutelare le famiglie e le imprese, dobbiamo essere consapevoli

sul lavoro e sulle imprese siamo stati in grado di prevenirli e governarli. Anche coloro che hanno tentato di accarezzare la protesta per ragioni di consenso e di propaganda non hanno trovato spazio. Molta di questa responsabilità sta nella misura e nella capacità che abbiamo avuto di tutelare il lavoro e quando parlo del lavoro parlo di tutto il lavoro. Abbiamo affrontato strategie inedite anche sul lavoro autonomo e sulle partite IVA. Non sarà ancora completo, ma abbiamo introdotto elementi di universalità nel sostegno al reddito, delle partite IVA e del lavoro autonomo che prima non c'erano in questo Paese e non eravamo in grado nemmeno di sostenere e progettare. Quindi, sono state fatte scelte emergenziali, ma dentro questa legge di bilancio ci sono anche alcune misure fondamentali per definire l'identità di una visione futura di questo Paese. Noi vogliamo riconoscere tutto questo. Il Partito Democratico vuole riconoscere tutto questo, perché è il nostro abito naturale e abita la democrazia, abita l'identità stessa di questa sfida, abita la responsabilità che ci stiamo assumendo e che ci vogliamo continuare ad assumere di portare l'Italia fuori dalla crisi. Lo ha Lo ha detto bene il senatore Zanda e io sono molto d'accordo, nel pieno richiamo del dettato costituzionale: noi dobbiamo considerare emergenziale l'*iter* parlamentare che i diversi decreti-legge hanno adottato. La forza e l'autorevolezza della politica sta anche nella capacità di questo Parlamento di riconoscere una condizione emergenziale e di non considerarla come qualcosa di naturale.

non avremmo avuto le condizioni per poter convertire una quantità così rilevante di decreti-legge economici come quella che il Governo ha introdotto. Dobbiamo riconoscerlo. un tradimento del dettato costituzionale; lo sarebbe e lo diventerebbe se noi consolidassimo una fase emergenziale in una fase naturale. Ma questo Parlamento e la politica devono avere l'autorevolezza di ritornare pienamente nel solco delle regole democratiche, ovviamente il senatore Zanda ha brillantemente indicato. Però ora siamo in una condizione emergenziale e dobbiamo tra di noi riconoscerlo. Ho ascoltato il rumore e il frastuono delle opposizioni, che, quando non hanno proposte, ritornano nella retorica della frammentazione, dell'acquisizione di banche, del conflitto con l'immigrazione. Siamo in un'altra stagione, è un'altra fase, c'è un volto nuovo dell'Europa. L'Europa ci mette in sicurezza, altro che acquisizione di banche. Senza le politiche monetarie della Banca centrale europea non avremmo avuto nessuna condizione per riportare lo *spread* a 111, da 270 di marzo, e per gestire un debito

Senza la sospensione del Patto di stabilità e senza iniziative europee tutto questo non sarebbe stato possibile. Oggi abbiamo questa nuova responsabilità di fronte a noi. Riconosciamo i limiti, ma dobbiamo anche avere un'ambizione grande. Avremo di fronte a noi la più grande opportunità per progettare il nostro futuro; la sfida nuova di questa maggioranza, oggi, è riconoscere queste priorità. Mi voglio soffermare su tre elementi fondamentali, che in parte sono abbozzati anche nella legge di bilancio. Abbiamo introdotto l'assegno universale sui figli: è la prima misura utile per rilanciare la famiglia e per togliere discriminazioni tra lavoro e lavoro autonomo. Soprattutto, è la prima iniziativa utile per correggere un insostenibile tasso di natalità, che ci spinge lontano dalle aree più virtuose del mondo. mondo. Rendere trasversali le politiche di genere significa correggere limiti strutturali, perché il tasso di occupazione femminile in questo Paese non può rimanere a questi livelli, se vogliamo costruire un futuro economico all'Italia. Questo lo dobbiamo rivendicare. Di fronte a noi ci sono sfide nuove; c'è bisogno di una visione. Non abbiamo bisogno di centinaia di progetti. Voglio partire da uno di essi, che secondo me è ancora trascurato e che invece va valorizzato: parlo della sanità. Se stiamo affermando che la prima misura economica consiste nel garantire il diritto alla salute ai nostri cittadini e dunque deve consistere nell'assicurare a loro e alle generazioni che verranno una protezione di fronte a nuove pandemie, noi dobbiamo avere un'accelerazione. Non mi interessa discutere per il momento della quantità di risorse; vorrei discutere di come ricostruiamo il volto della medicina territoriale, di come mettiamo in sicurezza i territori, di come siamo in grado di garantire i servizi ai cittadini. *(Applausi)*. Discutiamo prima di questo, altrimenti tutto ciò non ha senso nel rapporto con la nostra comunità. Questo vale anche per la digitalizzazione e per la riconversione in chiave ecologica della nostra economia. Su questi punti serve un'accelerazione; il Partito Democratico ne è consapevole, ha le sue proposte e mantiene la propria identità nella responsabilità di portare l'Italia fuori dalla crisi.

sento, in questo momento, di dover dedicare il nostro intervento al Presidente del Consiglio, che sta parlando in contemporanea con noi. *(Applausi)*. facendo la sua conferenza stampa di fine anno, nel posto giusto al momento giusto. In fondo, chi siamo noi? Noi siamo solo il Senato della Repubblica! che cosa stiamo facendo di importante? Stiamo solo approvando una legge di bilancio che non ci è neanche stato concesso di leggere! È giusto che il Presidente del Consiglio sia dov'è. Abbiamo sbagliato noi. Non abbiamo chiesto la diretta televisiva. Lo sanno tutti: no telecamere, no Conte!

Io non credo di poter fare lo stesso. Non credo di poter essere così veemente. Non credo di potermi spingere così avanti. Vorrei, però, a nome del mio Gruppo parlamentare, dire la mia, non solamente su questa legge di bilancio, ma sul modo in cui questa fase è stata affrontata. Noi stiamo vivendo una fase

la vostra incapacità di ammettere i vostri errori e dire che avete sbagliato, per la vostra incapacità di vedere il mondo reale. Ma voi le vedete quelle 390.000 imprese che stanno sparendo, che, anzi, sono già sparite? Quelle 390.000 imprese che hanno spento le luci per sempre? Li vedete quei 5 milioni e mezzo di poveri, ma poveri veri, di cui 2 milioni poveri da Covid-19? milioni di persone hanno visto precipitare drammaticamente il loro tenore di vita. E sapete chi sono? Gli artigiani e i commercianti, quelle partite IVA, quegli imprenditori, che vi stanno chiedendo da tanto tempo di essere aiutati, ma non con i DPCM, con gli Stati Generali,

e nei vostri mirabili interventi di opposizione, che però, mi sembra di capire, non esiteranno un voto contrario alla manovra. Tutto questo, in che modo può servire a un Paese allo stremo? A un Paese che sta veramente chiudendo le luci delle proprie fabbriche? Un Paese che sta chiudendo la porta dei negozi con la paura di non riaprirla più? più? Dietro quei banconi, dentro quelle cucine, ci sono delle vite, delle passioni, delle famiglie, delle storie. Costoro sono, con la loro creatività, con il loro sacrificio con la loro capacità di rialzarsi sempre, sono l'unica speranza di far rialzare l'Italia, se noi li aiuteremo. *(Applausi)*. Noi ci abbiamo provato. Abbiamo costretto la maggioranza ad approvare una decontribuzione delle partite IVA, una decontribuzione che è poca cosa. Come è poca cosa l'incentivazione dei trasporti; come è poca cosa la valorizzazione della disabilità nelle scuole paritarie; come è poca cosa l'*automotive*; come è poca cosa quanto abbiamo dato a medici e infermieri, che meritano tanto di più; come poca cosa è quanto abbiamo dato alle Forze dell'ordine. È poca cosa e noi chiediamo scusa per voi, per non avere fatto di più. Perché voi non siete capaci di chiedere scusa. Non siete capaci di ammettere i vostri errori e con una mano date uno e con l'altra mano prendete dieci. Avete decontribuito 3.500 euro per le partite IVA e dal primo gennaio fate partire 31 milioni di atti dell'Agenzia delle entrate *(Applausi)* - cartelle, accertamenti e avvisi che colpiranno il cuore produttivo di questo Paese, quelli che vi dicevo prima, quelli che tengono in piedi l'Italia, perché non siamo noi a tenere in piedi l'Italia, sono loro e noi li dobbiamo rappresentare ed aiutare. Questa è la nostra funzione, non fare finta di non vederli, non dire che la formula Italia è la migliore del mondo, non dire che va tutto bene, non fare inutili conferenze stampa autocelebrative mentre il Paese soffre. *(Applausi)*. Tutto questo non serve a niente, serve solo a prendere in giro il Paese e noi non lo vogliamo fare. Noi crediamo a quanto abbiamo fatto, siamo convinti che il nostro Paese abbia una grande opportunità, se riusciremo a dirci la verità, se riusciremo a farci dire la verità da voi. Per esempio, che cosa succederà il 7 gennaio? Le scuole

strumenti e mezzi di comunicazione e c'è un mondo reale che è quello che il Paese conosce molto bene. Cosa succederà? I nostri ristoratori, i nostri esercenti, i nostri impianti sciistici riusciranno a riaprire?

per un imprenditore è il peggiore dei mali. Non poter programmare, non poter sapere se deve fare contratti, se deve chiedere qualcosa ai fornitori, come programmare i propri bilanci futuri; non si può vivere di incertezze. Che cosa succederà? Riapriranno? Rimarranno chiusi? Guardate,

e bisogna fare un anno fiscale bianco. Basta, non possono pagare le tasse con i soldi che non hanno. *(Applausi)*. Noi lo esigiamo. Lo pretendiamo. E poi condono per chi non ce la fa. Sì, condono. Scandisco queste parole: anno fiscale bianco e condono per chi non ce la fa. *(Applausi)*. Questo è l'unico modo per risollevare il Paese. Altrimenti quei negozi chiusi, quelle fabbriche vuote, quelle saracinesche abbassate, non si rialzeranno mai più. Vaccini,

tutta Europa sta vaccinando come se non ci fosse un domani e noi facciamo vaccinazioni simboliche? *(Applausi)*. Che cosa vuol dire simboliche? Perché i nostri camioncini si fermano nella neve e gli altri no? Per quale motivo il commissario Arcuri ritiene di poter dire che non vuole rispondere a questa domanda? Comodo. *(Applausi)*. E io non voglio venire a lavorare. Il commissario Arcuri dovrà spiegarci il senso del suo simbolismo nei ritardi e nelle sue siringhe costosissime, che sembrano peraltro assolutamente inutili. Signori, questo non è uno scherzo. ogni giorno che passa è un ulteriore sacrificio di vite umane e noi non ce lo possiamo permettere. *(Applausi)*. Noi non siamo quelli che hanno fatto meglio di tutti; noi siamo quelli che hanno pagato più di tutti in termini purtroppo di morti per numero di abitanti e di crollo del PIL, come avete ricordato tutti. Non possiamo permetterci di pagare ancora. Next generation EU, meglio detto *recovery plan*; ve ne siete accorti anche voi, con i vostri interventi di maggioranza barra opposizione che sono numeri a capocchia, che sono i numeri del lotto quelli che avete messo in questo documento. *(Applausi).* Non è possibile. Lo ha detto persino il Ministro dell'economia, lo ha detto il commissario Gentiloni, lo hanno detto tutti. Ricordate quando dissi per la prima volta in quest'Aula che eravamo in ritardo?

il Presidente del Consiglio ci rispose: è una *fake news*. Adesso la *fake news* la diffonde anche il ministro Gualtieri. *(Applausi)*. Complimenti, almeno siete coerenti, dite tutti la stessa cosa. cosa. Vi dico due cose: il *recovery plan* non è la manna dal cielo, non è una cambiale che l'Italia presenta allo sconto e viene pagata pronto cassa: no, è la prova del nove della capacità di governare e di mettere a terra un vero sistema Paese che rappresenti le grandi, vere energie che l'Italia può produrre. *(Applausi)*. O così o si muore, anzi muoiono i nostri figli e i nostri nipoti di miseria, anche se questo ad alcuni può piacere. Signor Presidente, scriveva Oriana Fallaci che l'abitudine è la più infame delle malattie scriveva Oriana Fallaci che l'abitudine è la più infame delle malattie perché ci fa accettare qualsiasi disgrazia. Noi invece non ci abitueremo mai a voi né alle vostre disgraziate ricette, perché combatteremo sempre per le cose in cui crediamo, e noi crediamo nell'Italia e negli italiani, e crediamo fortemente che l'Italia si meriti un futuro all'altezza del suo straordinario passato. Per tutti questi motivi, noi voteremo no, no e no a questa miope, inutile, futile e tardiva legge di bilancio.

non ci stupisce, perché è parente stretto, ad esempio, di quel disprezzo che dimostrò per la cultura quando parlò di artisti che ci fanno divertire, come un monarca, come un sovrano del Medioevo. *(Applausi)*. Forse considera anche noi dei giullari, ma lasciamo perdere. L'ultima volta l'ho presa un po' larga; questa volta - me ne scuso - la prenderò larghissima e sarò anche un po' noiosetto. Vi dirò delle cifre, perché occorrerà anche mettere agli atti queste cifre, e alla fine dell'anno, cui ci siamo ridotti con la legge di bilancio, mi sembra un'ottima occasione simbolica per tirare una riga. Parto dal 28 giugno 1914, quando Gavrilo Princip assassinò l'arciduca Francesco Ferdinando, con le conseguenze che ricorderete. Mi limito a dirvi un dettaglio: il PIL italiano quell'anno fece un tuffo del meno 5,4 Ci vollero dieci anni perché il valore del 1913 venisse raggiunto e recuperato nel 1923, dopo aver toccato nel 1915 un minimo di 115 miliardi. In dieci anni recuperammo. Seconda puntata. In un afflato europeista, il 1° settembre 1939 la Germania invase la Polonia, perseguendo a modo suo - che nel frattempo è cambiato nelle forme, ma non nella sostanza, come vedremo - l'obiettivo di una unificazione del Continente, a suo uso e consumo. Quello che accadde dopo ce lo ricordiamo tutti, e anche qui mi limito a un dettaglio. Il PIL italiano nel 1939 crebbe di un gagliardo 6,3 per cento, ma poi le cose cambiarono per ovvi motivi, e si giunse a un minimo di 107 miliardi nel 1945 (quasi la metà). Anche in questo caso, però, bastarono dieci anni per raggiungere e superare il livello di partenza: nel 1949 il PIL italiano arrivò 201 miliardi. ci avviciniamo ad oggi. Nel 2007 scoppiò negli Stati Uniti quella crisi finanziaria che poi raggiunse la sua fase acuta, come ricordiamo, il 15 settembre 2008, quando Lehman Brothers portò i libri in tribunale. Nel 2007, il nostro PIL era di 1.795 miliardi. Qui però devo deludere i miei amici progressisti, quelli che a scuola, quando la professoressa spiegava Leopardi, erano un po' distratti: nonostante le magnifiche sorti e progressive, questa volta dieci anni non sono bastati per recuperare. Nel 2017 eravamo ancora del 5 per cento sotto il livello del 2007, a 1.704 miliardi, anni dopo, nel 2019, l'anno scorso - un anno che, guardato con gli occhi di oggi, ci sembra quasi normale - eravamo ancora sotto del 4 per cento, a 1.726 miliardi. Quanto ci sarebbe voluto, nel 2019, a tornare al livello pre-crisi? Al tasso medio di crescita che l'Italia ha registrato fra il 1999 e il 2019, pari allo 0,45 per cento, si sarebbe dovuto aspettare il 2028, cioè ventun anni, più del doppio di quanto era occorso per recuperare in occasione degli eventi bellici del XX secolo, per raggiungere e superare il livello pre-crisi del 1997. Vengo al punto. Quando qui oggi qualcuno si intenerisce sui cosiddetti errori del passato, sull'austerità che - signora mia - fa tanto male alla crescita, la mia sensazione è che non sappia proprio di che cosa si sta parlando. Questi dati lo illustrano: le regole europee hanno raddoppiato il nostro tempo di recupero e prolungato le nostre crisi, di qualsiasi natura, portandole da dieci a vent'anni.

però, seguendo il vostro discorso, quello che ci ha bloccati, la malattia, non è il Covid, ma, dal 1997, l'adozione del Patto di stabilità e crescita, quindi un'altra malattia: l'austerità europea, la *governance* economica europea, il semestre europeo (sì, proprio lo stesso che dovrà gestire i soldi del *recovery).* Come potrà andare a finire? Ora voi siete tutti costretti a dire quanto noi dicevamo nel 2012, cioè che l'austerità è un errore. La mia domanda è se c'era bisogno del Covid per accorgersene, quindi per sospendere le regole. La risposta è nei dati che vi ho fornito ed è no. Chi voleva vederlo lo avrebbe già potuto vedere: era già chiaro che qualcosa non andava. Adesso, però, ragioniamo sulle conseguenze del Covid, *pro futuro*. Le ultime previsioni della Banca d'Italia dicono che quest'anno faremo il meno 9 per cento, un buco di 155 miliardi, che ci porterà intorno a 1.571 miliardi, cioè torneremo ai valori precedenti alla malattia (perché nel 1998 il PIL italiano era più o meno lì, a 1.574 miliardi) e poi ci sarà il rimbalzo. Certo, il rimbalzo doveva essere del 6 per cento e oggi la Banca d'Italia lo quota al 3,5, ma solo

che ora le regole sono sospese e abbiamo una pioggia di miliardi, che è una grande opportunità, quindi dobbiamo fare presto. Mai sentita questa esortazione? Ragioniamo sulla sospensione. Perché le regole venissero sospese non è bastato che danneggiassero il nostro Paese al punto da raddoppiare la durata della sua crisi, ma è dovuto succedere qualcosa che oltre a noi mettesse in difficoltà la potenza egemone, quella stessa che le regole, i trattati e i contratti li applica e disapplica a suo piacimento, nella vostra indifferenza. Voi, intanto, avete alimentato, con i vostri "intellettuali" e i vostri *media*, una narrazione abietta, che colpevolizzava il popolo italiano per un fallimento che altro non era che la leale adesione a regole assurde di cui oggi dovete riconoscere l'assurdità. E gli altri intanto come si regolavano? Vi faccio un esempio. Quando la Germania, a giugno di quest'anno, ha deciso di procedere indennizzando i costi fissi delle imprese, non ha chiesto permessi: l'autorizzazione europea è arrivata dopo, a ottobre, con la quarta modifica del quadro temporaneo di aiuti, ma intanto il Governo tedesco aveva agito. Non lo critichiamo per questo, sareste voi a doverlo fare, voi che siete così babbalei da credere all'Europa della solidarietà e voi che continuate a credere che la difesa dell'interesse nazionale sia deprecabile, perché il bene del tutto per voi giustifica sempre il male delle parti, siano la Grecia o - peggio ancora - la vostra parte, l'Italia. Vi faccio un altro esempio. Avete letto l'allegato alla COM n. 4192 del 2020, la decisione della Commissione che stabilisce la strategia vaccinale europea? L'articolo 7, rubricato «Obbligo di non negoziare separatamente», recita: «Firmando questo accordo gli Stati membri confermano la loro partecipazione alla procedura e acconsentono a non lanciare procedure nazionali per anticipare l'acquisto di vaccini dagli stessi produttori».

diamo torto invece a chi ciancia di Europa cambiata e di grande prova di solidarietà, senza voler affrontare il nodo della questione, che non è la sospensione, ma il totale ripensamento delle regole. È tutto in questa storia di ordinaria subalternità il motivo per cui gli italiani che noi ci onoriamo di rappresentare non hanno fiducia in voi. per il vostro rifiuto di confrontarvi con la realtà, per la vostra incapacità di rivendicare pari dignità per il nostro Paese e per l'aperto disprezzo che avete dimostrato verso di loro, verso gli italiani. Anziché parlare di miliardi che in gran parte non ci sono - e che, se ci saranno, dovranno comunque essere restituiti, dopo essere stati gestiti secondo le regole che hanno distrutto la nostra economia - e ringhiare come cani attorno a un osso per spartirvi il prestito che arriverà, lasciando chiudere le aziende e fallire le imprese che poi dovranno ripagarlo (cosa che ben vi guardate dal dire), dovreste porvi qui e in Europa l'unica domanda urgente che abbia senso porsi oggi: come cambiare la *governance* economica europea e cosa fare se questo dovesse rivelarsi impossibile. Tale operazione di verità, però, vi è preclusa per motivi non etici, ma etologici. Preferite continuare a tirare a campare, di rinvio in rinvio: meglio un sussidio domani che la dignità oggi!

Senatore Bagnai, sto controllando una sua espressione con riferimento a un paragone tra la situazione della Germania e della Polonia,

Potrei aggiungere «finalmente» oppure potrei cercare comunque qualcosa di positivo in un anno certamente complicato per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo intero. Preferisco questa seconda opzione, perché solo analizzando ciò che è successo potremo lavorare al meglio per costruire l'Italia del domani e questo lo voglio sottolineare soprattutto per i colleghi dell'opposizione, che sono sempre bravi solo a criticare, ma mai a collaborare. *(Applausi)*. In questi dodici mesi complessi, anche per quanto riguarda il lavoro parlamentare, ho avuto l'opportunità e l'onore di essere Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione bilancio.

colleghi, facciamo parlare la senatrice Accoto. Non c'è bisogno di fischiare. Ognuno dice quello che vuole.

un ruolo importante, con molte responsabilità, nel quale ho dato tutta me stessa per offrire le risposte che tutti i cittadini si aspettano nei provvedimenti che licenziamo come Parlamento. Per questo, la narrazione del presente disegno di legge di bilancio non può essere decontestualizzata dal lavoro di un intero anno e ancor di più dai provvedimenti di questi ultimi mesi. Credo che questa manovra non sia stata valorizzata abbastanza per quanto di buono vi è contenuto - desidero proprio sottolinearlo - forse per le tempistiche che ha avuto il suo *iter* parlamentare; incastrata com'era tra provvedimenti emergenziali, non le si è riconosciuta l'innovatività che invece ha in molti dei suoi interventi. Ha un impianto chiaro, strutturato attorno a quattro grandi pilastri, per dare una spinta decisiva alla ripresa: parlo di sanità, scuola e digitalizzazione, imprese e lavoro, famiglia e e politiche sociali. Si tratta di 40 miliardi di euro che si aggiungono agli oltre 100 già stanziati nel corso dell'anno per far fronte allo sforzo economico senza precedenti sostenuto a partire da marzo. La manovra agisce, da un lato, sul fronte emergenziale con provvedimenti come la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione; misure che - lo ricordiamo - ci hanno consentito di scongiurare circa 600.000 licenziamenti. Abbiamo inoltre valorizzato lo straordinario lavoro dei nostri medici ed infermieri, con ulteriori risorse destinate a retribuire le dovute indennità e, al contempo, a potenziare l'assistenza territoriale. Un altro tassello fondamentale in tale direzione è dato dall'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture e dei presidi territoriali della Sanità militare che, con dedizione ed impegno, ha dato un grande contributo nell'affrontare l'emergenza sanitaria, al fine di evitare il sovraccarico dei nostri ospedali. Dall'altro lato, invece, si è puntato tutto sull'innovazione del Paese, per consolidare la ripresa della produzione che - giova ricordarlo - nel terzo trimestre dell'anno ha raggiunto un aumento del 16,1 per cento rispetto alla stima prevista (più 11,2 Tutto questo grazie a misure ambiziose, come il Piano nazionale transizione 4.0, gli ulteriori contributi previsti per le piccole e medie imprese

Ma non solo. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre avuto a cuore il futuro dei lavoratori e la loro formazione. Per questo destiniamo 500 milioni alle politiche attive del lavoro. Per incentivare le assunzioni e la creazione di lavoro, crediamo infatti che sia necessario intervenire sulla riqualificazione dei lavoratori e sulla riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. Per questo, con la decontribuzione integrale per l'assunzione di giovani *under* 35, aiutiamo le nuove generazioni ad inserirsi nel mondo del lavoro. Sarà lo Stato a farsi carico fino al 2023 del pagamento del 100 per cento dei contributi totali che un'impresa deve sostenere quando decide di assumere un lavoratore. *(Applausi)*. Infine, permettetemi anche di sottolineare come ci siamo battuti per la proroga del superbonus al Quest'agevolazione è stata fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle e, con il voto in Commissione bilancio alla Camera, è stata estesa per tutti fino al mese di giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici condominiali che a giugno abbiano realizzato almeno il 60 per riforme innovative per un'Italia che non lascia nulla di intentato per proiettarsi nei prossimi decenni; una narrazione politica coraggiosa (quasi avventurosa, sicuramente elettrizzante), che potrei accomunare ai contorni di una grande trilogia cinematografica.

e tornare alla propria vita normale. Ad esempio, gli ultimi decreti - mi riferisco alla quadrilogia del ristoro - possono essere considerati *sequel* di un primo grande film, ma riescono a essere quasi migliori dell'opera prima e costituire, anche insieme a questa manovra di bilancio, un corpo unico e indivisibile. Queste opere hanno avuto un grande regista, che voglio ringraziare personalmente: il presidente Giuseppe Conte. *(Applausi)*. Egli ha saputo essere collante per tutta la maggioranza e, con il suo spirito risoluto, ha saputo procedere con estrema convinzione nel suo lavoro, molto complicato, di trovare risposte a una crisi mai vista prima d'ora. Dove c'è un *film*, ci sono gli spettatori. Chi è il nostro pubblico? Ovviamente sono tutti gli italiani (non solo le persone, ma anche le aziende, gli imprenditori e i liberi professionisti),

Voglio dirvi, colleghi, che quel coraggio di cui parlo l'ho visto in questi mesi in tutti gli attori che, insieme a me, hanno partecipato a tutte le riunioni dei Capigruppo con il Governo. Nessuno ha mai gettato la spugna, né si è mai limitato a fare il minimo sindacale. Se un buon attore fa un'interpretazione scialba, può inficiare tutto il risultato finale di un *film.* Per questo, posso confermare che tutti, fino a oggi, hanno dato il loro meglio (o, almeno, quasi tutti). Mi viene da sorridere, pensando a quale *film* avrebbe potuto girare qualche collega senatore che siede dall'altra parte dell'emiciclo: mi viene in mente un qualcosa di simile a un *trash movie*. A questo abbiamo assistito, fortunatamente per meno di un anno: un *film* che voleva scimmiottare Clint Eastwood nell'ispettore Callaghan. Il problema è che, invece dei criminali, ci si è intestarditi nel voler forzare le prerogative del Ministero dell'interno e far finta che il diritto internazionale non esistesse. colleghi, concludo il mio intervento con l'auspicio che molte norme innovative contenute in questa manovra di bilancio non si esauriscano nel 2021. Anche ad alcuni colleghi di maggioranza voglio ricordare che chi non ha il coraggio di scalare una montagna non può certamente cadere, ma chi rimane in pianura mestamente vivrà una vita priva di emozioni, passione e gioia. Lasciatemi dire che nel MoVimento 5 Stelle non viviamo in questo modo. Pertanto, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al disegno di legge di bilancio.

cortesia? Stiamo varando la legge più importante dell'anno e lo stiamo facendo in un giorno.

Volete essere europeisti e campioni di europeismo, ma pigliate sberle. La Germania, sul piano vaccinale, ancora una volta, vi ha ricordato le regole del gioco: l'Europa è loro, è cosa loro. La Germania fa quello che vuole? Italexit è qui a dirvi: bene, ognuno pensi da Stato sovrano, libero e autonomo. Brexit è la vittoria dei britannici. Basta con questa euroipnosi dannosa, drammaticamente dannosa. La Germania ha fatto quello che voleva sui vaccini esattamente come l'ha fatto con la ripartizione dei migranti e con il *surplus* della bilancia commerciale, in continua violazione delle regole. Lo ha fatto salvando le proprie banche e coprendo i suoi Paesi alleati, che sono paradisi fiscali. Oggi ci proponete l'ennesimo esercizio artificiale di contabilità, altro che ripartenza economica: è la quarta versione di "promettopoli", che funziona un pochino dentro questo specchio deformante dei Palazzi, ma fuori non funziona per niente, dove c'è un Paese che in silenzio sta male, e attenti a quello che cova. E voi cosa fate? State ancora dietro ai Benetton, che maramaldeggiano sul creato da Conte e sostenuto dal ministro Patuanelli, il ministro amico del giaguaro. Ci sono stati 44 morti a Genova e non avete revocato un tubo! Del resto, state facendo ingrassare le multinazionali; cosa vi interessa delle piccole e medie imprese? State cercando di regalare quella Monte dei Paschi di Siena su cui tutti gli italiani hanno dovuto mettere i soldi, in modo da poter controllare una banca. Arrivate con una manovra zeppa di *bonus*. Ma lo volete capire che per acciuffare un *bonus* bisogna superare una gincana di scartoffie? Alla faccia delle semplificazioni. Parlate del Covid con linguaggio di guerra e poi volete ricostruire senza soldi e senza idee. Dovevate resettare alcune voci fiscali e abbattere il costo del lavoro, gli oneri di sistema nelle bollette e le accise sulla benzina dovevate promuovere un giubileo sulle sofferenze bancarie: e invece ora, dalla vostra cara Europa, arriva un'altra vergognosa ingiustizia su chi è sul filo del conto corrente in banca. Tutto questo costa? Certo che costa, e tanto. Ma chi paga? Lo Stato, con la sua moneta sovrana. Sapete cos'ha fatto adesso il Governo giapponese? Un piano da quasi 840 miliardi di euro. È il terzo anno di fila che il Giappone approva manovre da oltre 100.000 miliardi di yen e lo fa perché ha moneta sovrana ed è proprietario del proprio debito pubblico, del quale non ha paura. Tenetevi dunque le regole idiote dell'Europa. Italexit se ne vuole andare e non ha paura, perché noi siamo l'Italia.

Signor Presidente, gentili colleghi, come previsto, siamo giunti all'ennesimo voto di fiducia alla cieca. È vero che sta diventando una prassi, una prassi incostituzionale, ma quest'anno l'emergenza Covid ha anche peggiorato la situazione. Ne abbiamo prova dalla pioggia di decreti che una Camera a turno esamina e l'altra può solo ratificare, solo ratificare, senza intervenire. Si tratta di una prassi confusionaria, alla quale quest'anno si è anche aggiunta l'invenzione dei decreti ristori,

giustamente a reclamare dinanzi alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzioni e affermando che il metodo di approvazione semplificata e contratta nel tempo della legge di bilancio del 2019 violava, come poi la Corte ha confermato, le prerogative di ciascun singolo senatore. Allora, come ora, non era stato possibile esaminare il provvedimento, né discutere gli emendamenti. Oggi, pur mutando le circostanze, la sostanza - senatore Errani, mi rivolgo anche a lei - non muta affatto. Questa prassi è incostituzionale e sbagliata e depriva non soltanto il singolo parlamentare, ma il Parlamento e, in definitiva, anche lo stesso Presidente della Repubblica del dovere di esaminare *funditus* la legge di bilancio, la legge più importante dello Stato. L'articolo 73 della Costituzione, infatti, riconosce al Capo dello Stato un periodo fino a un mese

del dovere di correggere i propri errori. Per questi motivi di metodo e per tanti altri di merito lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio ha definito questa legge di bilancio un insieme confuso e un coacervo indistinto senza disegno. Per tutti questi motivi,

ma le diamo a supplenti, per giunta non abilitati. C'è un'illogicità nella gestione del personale che non ha precedenti.

Vi pregherei di non creare assembramenti in Aula, colleghi, vedo troppi ammassamenti.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento,

il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Nencini.

Marinello,

naturalmente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

ha posto la questione di fiducia:

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge.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

Questa è una grande vittoria non solo dei parlamentari della Lega, che fortemente hanno sostenuto e supportato l'Alta velocità, ma del Paese intero. La non partecipazione al voto dei 5 Stelle sottolinea ancora di più la bipolarità di questo partito e dei suoi componenti, ecologisti a fasi alterne favorevoli all'uso indiscriminato dei monopattini in città, ma ostili a un'opera che comporterà una diminuzione di gas serra pari all'anidride carbonica prodotta da una città di 300.000 abitanti, come Catania o Bari. Bari. Chiedo un moto d'orgoglio al ministro Lamorgese per tutelare i lavoratori del cantiere e le Forze dell'ordine che ne garantiscono la sicurezza. Suggerisco l'istituzione di un blocco, per motivi di sicurezza, del sentiero gallo-romano, agli anarco-insurrezionalisti che periodicamente attaccano il cantiere. Potrebbe essere all'altezza del campo sportivo di Giaglione. Questo onde evitare situazioni oltremodo disdicevoli per un Paese evoluto quale io credo sia l'Italia, come quella occorsa il 13 dicembre scorso, quando un poliziotto, ferito dai poco pacifici manifestanti, è stato portato in ospedale non da un'ambulanza ma da una carriola, prima, e da un'auto privata, poi. Economicamente parlando, la ricaduta sarà pressoché immediata dal momento che arriveranno in Provincia di Torino 90 milioni di euro per le opere compensative ai Comuni che hanno subito disagi e che si sommeranno agli 8.000 posti di lavoro che il cantiere porterà sul territorio. In un momento storico economico come quell'attuale, massacrato dalla pandemia, le opere infrastrutturali sono il volano ideale per far ripartire l'economia. Noi piemontesi siamo stufi di non essere considerati. Non vogliamo vivere di sussidi. Vogliamo continuare a lavorare e, anche grazie alla TAV, il Piemonte potrà essere protagonista del rilancio economico dell'Italia *post* Covid. *(Applausi)*.

*(M5S)*. Signor Presidente, questo è stato un anno molto difficile e, anche in quest'Aula, non sono mancati momenti di scontro, parole dure, situazioni anche facilmente giustificabili, pensando alla politica come tanti di noi l'hanno pensata prima di candidarsi in tale ruolo. Ci sono stati anche momenti di scontro duro, ma si è sempre trattato di situazioni tra pari, tra persone che hanno la capacità di difendersi sia legalmente sia dialetticamente. Purtroppo, in questa fase di continua tensione, alcuni personaggi del mondo della comunicazione, e purtroppo anche delle istituzioni, si sono invece distinti per una pratica che personalmente ritengo assolutamente fastidiosa, cioè quella di offendere tirando in ballo intere categorie. È successo a tanti di noi, di tutti gli schieramenti, ed è successo l'altro giorno al sindaco di Roma Virginia Raggi, nel momento in cui il collega - chiamiamolo così - Vittorio Sgarbi della Camera,

di prospezione e di coltivazione di idrocarburi, così come stabilito dalla legge n. 12 del 2019, nell'attesa della realizzazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). Signor Presidente, ogni legge ha il suo scopo: quello della legge in questione è di favorire la sostenibilità ambientale, annullare l'impatto delle attività *upstream* e accompagnare il processo di decarbonizzazione. si individuano più facilmente le aree idonee per le attività estrattive, tenendo conto di alcuni fattori molto importanti, come le caratteristiche territoriali, sociali, economiche, urbanistiche e morfologiche, nonché dell'impatto sull'ecosistema; stabilendo una volta per tutte in maniera chiara e nitida i criteri, vale a dire i tempi e i modi di ripristino di quelle aree, quando verranno dismessi gli impianti; in pratica, tutto ciò che non è stato fatto in Basilicata negli ultimi vent'anni. Ricordo che la Basilicata è un territorio interessato per il 90 per cento da richieste di permessi di ricerca, prospezione e coltivazione questa legge interessa ai cittadini e anche molto, perché la tutela ambientale riguarda la tutela della propria salute e anche della propria economia.

che stanno chiudendo a causa della crisi energetica, sanitaria ed economica derivante da Coronavirus, ma quante ne abbiamo contate e ne conteremo, soprattutto nel settore agricolo, che chiudono i battenti a causa dell'inquinamento nel proprio territorio? È tutta una catena. Funziona così: chiude un'azienda, vanno via persone, chiudono altri esercizi commerciali di quel territorio e arriva una desertificazione sociale. È il fenomeno dello spopolamento. In Basilicata esistono pozzi di petrolio che insistono su falde acquifere a ridosso di ospedali, vicino invasi la cui acqua serve per l'irrigazione dei campi agricoli, oltre a pozzi di reiniezione. In conclusione,

fornire ai cittadini lucani uno strumento idoneo affinché possano dire finalmente la loro sul tema del petrolio.

sulla strada sulla quale si affacciava il suo ufficio presso Rocca Salimbeni, a Siena. Le numerose indagini aperte dai magistrati, nonostante il sequestro del suo telefonino dal quale vennero cancellate 300 *e-mail*, tra telefonate e messaggi che avrebbero fatto fatto piena luce su quella misteriosa morte, non hanno portato a nulla; mentre la più antica banca, fondata nel 1472 come Monte di pietà per dare aiuto alle classi disagiate della città, che durante i secoli era riuscita a resistere a guerre, carestie, pestilenze e terremoti, non è riuscita a resistere a una gestione sciagurata del credito e del risparmio, inghiottendo in un grande buco nero 60 miliardi di euro tra aumenti di capitale e distruzione di soldi pubblici e privati sborsati dagli azionisti. Oggi quella banca, in parte risanata coi fondi pubblici, rischia di essere regalata alla banca di Alessandro Profumo, quella Unicredit presieduta da un ex deputato ed ex Ministro dell'economia, in deroga a precise direttive europee

L'Italia ha ritardato per sette anni il recepimento di quella direttiva, con l'ultima versione predisposta dall'ex ministro Padoan, che prevedeva norme stringenti contro i conflitti di interesse dei banchieri da nominare, al comma 3 dell'articolo 24. Ebbene, il ministro Gualtieri,

Francesco Castiello purtroppo è ricoverato al Gemelli da un paio di giorni: facciamo a lui e a tutti gli ammalati di Covid-19

intesa come mancata conoscenza del sistema sanitario tutto, e non solo di quello calabrese, da parte di chi invece dovrebbe avere a cuore la salute come bene assoluto, secondo la nostra Costituzione alla storia della sanità calabrese aggiungiamo nuovi tasselli che, inquadrati sia nel pubblico che nel privato, dipingono un quadro organizzativo abbandonato a se stesso. Intervengo oggi per sottoporre all'attenzione del Senato il caso della clinica Sant'Anna Hospital di Catanzaro, un centro di riferimento per tutto il Sud Italia per la cardiochirurgia specialistica, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, che è al centro di una diatriba che, al di là dell'emergere di carenze, illegittimità e inchieste della magistratura, in cui riponiamo ampia fiducia e che devono continuare il loro corso, coinvolge non solo la *governance* della struttura, legittimata finanche da un'ordinanza del giudice per ma ovviamente i dipendenti e, soprattutto, tutti gli utenti, calabresi e non. Il mancato pagamento da parte dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catanzaro delle prestazioni regolarmente erogate, ammontante a circa 23 milioni di euro, e l'assenza di un confronto, attraverso la convocazione di un tavolo tecnico che aggiorni su quello che dovrà essere il futuro dell'ente di eccellenza della sanità calabrese, mettono la clinica nell'impossibilità di continuare a erogare diligentemente come ha sempre fatto i servizi di prestazione specialistica. Chiediamo dunque, per il centro di Sant'Anna, che rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla migrazione sanitaria, realizzando un attivo e non un passivo per la Regione, che il commissario *ad acta* intervenga con sollecitudine, deliberando un piano eccezionale di mantenimento dei servizi, da estendersi per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale. Ciò permetterebbe alla gestione manageriale di porre in essere, una volta per tutte, le misure necessarie

Per una volta, la burocrazia lasci il posto al buon senso e il commissario *ad acta*, se ha un senso che ci sia, agisca, affinché si possa permettere la ripresa delle attività in sospeso la necessaria cura dei cittadini affetti da patologie cardiologiche gravi e in attesa di una speranza.

con la sentenza di appello di ieri sulla vicenda delle mense di Lodi si è compiuto un atto di giustizia importante in questo Paese. Vorrei però porre una questione all'attenzione di quest'Assemblea: quando sollevammo il tema e interrogammo anche l'allora Ministro dell'istruzione, chiedendo un intervento sulla vicenda che purtroppo non fu posta in essere, ponemmo una questione politica. Ora è bene che la magistratura faccia il suo corso; c'è la divisione dei poteri e per fortuna in questo Paese c'è uno stato di diritto e viene e viene ripristinato un principio importante. È un peccato che l'amministrazione comunale di Lodi abbia resistito a questo e abbia anche speso molto denaro pubblico per niente, invece che prendere atto di un dato di fatto. Ma c'è un tema che è profondamente politico su cui vorrei che quest'Assemblea riflettesse. riflettesse. Quella decisione scellerata di trovare dei cavilli burocratici per impedire a bambine e bambini di partecipare al servizio di mensa, come un fatto normale e logico e di civiltà,

deve diventare un sentimento comune del Paese, che dovrebbe appartenere a tutte le forze politiche e chiudere un'era in cui abbiamo utilizzato il migrante come un nemico; un sentimento che dovrebbe riportare questo Paese ad essere nel mondo un alfiere di giustizia, civiltà, incontro e inclusione, come tra l'altro la nostra straordinaria storia ha sempre rappresentato. *(Applausi)*. Signor Presidente, ieri abbiamo avuto la notizia della condanna di dieci attivisti per la libertà di Hong Kong, per aver tentato di uscire dal Paese e di andare a Taiwan. Hong Kong è ormai diventata una prigione. Era uno dei

del 18 agosto 2020, in cui chiedevo conto del vergognoso voto di astensione dell'Italia quando alle Nazioni Unite si è trattato di condannare la legge sulla sicurezza di Hong Kong che sta creando ogni giorno dei danni e sta rendendo la Cina particolarmente aggressiva verso altri Paesi, tra cui l'Australia, nella sua politica espansionistica generale. Sollecito anche la risposta all'interrogazione

a cui sono stati sottratti quattro bambini con motivazioni ancora assai poco chiare. Orrore degli orrori, quei quattro ragazzi, tra i sei e i sedici anni, sono stati separati fra di loro,

Essendo l'ultimo intervento di quest'anno, colgo l'occasione, Presidente, per formulare a lei i migliori auguri per l'anno nuovo e, insieme a lei, a tutti i colleghi presenti e ai funzionari del Senato, rappresentati nel suo massimo vertice dal Segretario generale, nonché al rappresentante del Governo che è anche nostro collega.